non è riportato il contenuto delle interruzioni che ho fatto: esse sono state troppo vivaci e me ne dolgo con l'Assemblea e con lo stesso Presidente; mi dolgo del tono non particolarmente gentile con cui si è rivolto nei miei confronti, perché mi rendo conto delle difficoltà di gestire una seduta così complessa. Avendo fatto, tra gli altri mestieri in gioventù, anche quello di resocontista di Assemblea, non mi dolgo nemmeno del modo con cui sono state o non riportate le mie interruzioni, perché so bene in quali condizioni si svolge il lavoro del resocontista tanto più quando, come è giusto, dall'altra parte c'è il Presidente del Senato. Vorrei, però, precisare il mio pensiero al riguardo, perché è la prima volta che negli atti parlamentari - da quindici anni che sono senatore vengono riportate "*Vivaci proteste*"; come tutti i colleghi sanno, non c'era alcun insulto, ma il tentativo di fare una considerazione che oggi vorrei svolgere e che vorrei restasse agli atti. Non mi riferisco tanto alla questione dell'ammissibilità o meno del voto su un comunicato stampa. Ringrazio i colleghi, in particolare il presidente Matteoli, che, con la consueta sensibilità istituzionale, hanno colto il punto. Quello che volevo dire è che i giudizi sulle ammissibilità o sulle preclusioni fanno parte dei precedenti parlamentari perché, come è noto, il diritto parlamentare si interpreta alla luce dei precedenti. Quello che vorrei restasse agli atti - ripeto, non come critica o come ritorno sulla valutazione, ma perché fosse chiaro che ciò non costituisce un precedente, è che, a mio avviso, non può essere considerata ragione d'inammissibilità di una proposta di risoluzione - mi riferisco alle motivazioni date circa l'ammissibilità della proposta di risoluzione relativa a Vicenza - la circostanza che il Presidente del Consiglio abbia annunciato, sia pure in sede parlamentare, una certa decisione. In effetti, delle due motivazioni che il Presidente ha dato della inammissibilità, la prima, ovvero il fatto che non concernesse il tema oggetto della seduta, rientra alcuni colleghi hanno avuto un'opinione diversa - nei giusti rapporti tra Governo e Parlamento; a mio avviso, non vi può rientrare in alcun modo il fatto che il Presidente del Consiglio o il Governo, abbiano annunciato una certa decisione. Essendo quella del Parlamento funzione di indirizzo e di controllo è del tutto chiaro che, a mio avviso, è legittimo - ripeto, salva l'altra questione di ammissibilità - e quindi non può restare come precedente agli atti dell'Assemblea, che possa essere motivo di ammissibilità di una risoluzione o di un ordine del giorno la richiesta di uno o più parlamentari di chiedere al Governo di modificare una decisione, ancorché annunciata ufficialmente nelle diverse sedi. Direi, anzi, che fare questo è il sale della democrazia parlamentare.

Presidente, desidero scusarmi se ieri sera sono intervenuto in Aula senza la sua autorizzazione ed in modo alterato a causa anche della mancanza del microfono. Di fronte, però, all'atteggiamento di bullismo o di saccenza che il ministro D'Alema ha avuto nel voler ricordare all'Assemblea le prerogative di noi parlamentari, cioè la possibilità di ricorrere ad interrogazioni ed interpellanze, gradirei che lei usasse tutta la sua fermezza e le sue capacità di convincimento verso il Governo Prodi, quindi non solo verso il Presidente del Consiglio ma verso tutti i suoi Ministri, affinché vengano realmente rispettate le prerogative dei parlamentari, tra cui la prima sono proprio gli atti di sindacato ispettivo. Ho presentato una decina di interrogazioni, ho avuto risposta finora ad una interrogazione scritta dal vice ministro Minniti che, peraltro, rispetto ad una interrogazione molto chiara e precisa, ha risposto con parole del tutto prive di senso, ricordandomi la normativa che conosco bene su quella materia.

delle interrogazioni presentate. Se fosse così, credo che lei, a tutela del prestigio di quest'Assembla, debba ottenere un cambiamento di rotta dal Governo. Diversamente, le anticipo che farò ricorso anche al Capo dello Stato su questo argomento, in modo tale che egli, che è stato parlamentare e Presidente di una Camera, possa vedere di interporre non certo i suoi buoni uffici, ma piuttosto una dura risposta ad un Governo arrogante. ringrazio, senatore Paravia, io colgo il senso vero del suo invito. Capisco che ci sono ritardi, ma cercheremo di migliorare la situazione; l'impegno della Presidenza del Senato è assicurato.

rappresentante del Ministero dell'interno per riferire all'Aula. Voglio ringraziare il sottosegretario Rosato che, con assoluta sensibilità, ha accolto, appena possibile, il nostro invito

non solo per le due vittime che abbiamo constatato, ma anche per l'emergenza climatica che caratterizza questo periodo l'emergenza criminale connessa agli incendi che si sono sviluppati in tutto il Mezzogiorno del Paese. Per dare un dato simbolico che può rendere evidente l'emergenza che stiamo affrontando in questi giorni, che ieri mi auguro abbia avuto il suo apice, solo i centralini dei Vigili del fuoco hanno ricevuto 40.000 chiamate; nella giornata di ieri ci sono stati 2.000 interventi solo dei Vigili del fuoco per incendi boschivi e il COA, il dipartimento della Protezione civile, ha ricevuto 100 chiamate per le emergenze di tipo aereo. È corretto ricordare come in relazione all'annoso problema che si ripete degli incendi boschivi il Presidente del Consiglio dei Ministri, cui è affidato il compito di stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 luglio 2005, n. 152, l'avvio della campagna estiva, ha dettato indirizzi operativi per fronteggiare i rischi degli incendi boschivi per la stagione estiva 2007, inviando, come tutti gli anni, una nota alle Regioni e ai Ministri competenti in data 1° giugno 2007. In questa nota, si ricordava il rispetto delle competenze attribuite alle Regioni e alle Province autonome dalla legge quadro per gli incendi boschivi, la n. 353 del 2000, e della sinergia necessaria fra tutte le componenti deputate allo spegnimento, che il Presidente ha sottolineato con l'attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi. Il Presidente ha fatto appello alla necessità di un'azione congiunta tra le Regioni e tutte le autorità competenti. Credo sia utile ricordare come la legge n. 353 affida in maniera inequivocabile alle Regioni l'attività di previsione e prevenzione del rischio degli incendi boschivi, nonché la lotta attiva che comprende le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra e aerei. La medesima legge invece affida al Dipartimento di protezione civile il coordinamento sul territorio nazionale delle attività aeree di spegnimento mediante la gestione della flotta antincendio Di fatto, a partire dal 22 luglio, così come è sotto gli occhi di tutti, c'è stato un crescendo esponenziale del numero degli incendi e conseguentemente di interventi da parte dei Il 22 luglio abbiamo registrato 71 richieste d'intervento, il 24 luglio, come dicevo prima, 100 interventi. È possibile e utile fare un confronto con il 2003, un anno eccezionale rispetto alla crisi estiva, riconosciuto come l'anno più caldo e siccitoso degli ultimi cinquant'anni, eppure i picchi massimi giornalieri delle richieste non superarono nemmeno della metà quelli che abbiamo riscontrato negli ultimi giorni. Una delle zone dove più drammaticamente abbiamo riscontrato una situazione d'emergenza è stata quella della Puglia, dove si è verificata una grave situazione su cui mi soffermerei con maggiori dettagli più avanti, in cui abbiamo registrato anche i due deceduti, ma bisogna dire che gli incendi si sono sviluppati in tutte le Regioni del Centro e del Sud Italia, con particolare criticità in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, dove ancora oggi la situazione è preoccupante, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise e in Basilicata. Basilicata. Complessivamente la flotta aerea messa a disposizione per fronteggiare l'emergenza è stata tutta impegnata, con 13 Canadair, cinque elicotteri del Dipartimento della protezione civile, elicotteri del Corpo forestale dello Stato, due elicotteri dell'Esercito italiano messi a disposizione dal Ministero della difesa, così come tre elicotteri della Marina Militare e dieci elicotteri del Dipartimento dei Vigili del fuoco.

In particolare, poi, i Vigili del fuoco hanno spostato le loro colonne mobili dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Lazio, dalla Campania, dall'Emilia-Romagna e dalla Toscana verso le aree maggiormente colpite del Paese. del Paese. Tre eventi sono stati particolari per la loro gravità: il primo riguarda l'incidente occorso ad uno dei mezzi aerei del soccorso, in cui ha perso la vita il pilota del Canadair e un altro è in gravi condizioni, anche se al momento stabilizzate, e ci auguriamo veramente nelle prossime ore di avere buone notizie; il secondo è stato l'incendio di vaste proporzioni che ha colpito la zona di Vieste e Peschici, in provincia di Foggia, ed il terzo, ahimè, è la conferma che la maggior parte di questi incendi sono di natura dolosa. Rispetto all'incidente che ha coinvolto il Canadair, dobbiamo dire che questi uomini sono stati lungamente impegnati in giornate particolarmente intense, che il loro lavoro è particolarmente rischioso, ricordato, e che l'incidente è avvenuto durante un volo alla fine della giornata, con uno sgancio dell'acqua a circa 30 metri dal suolo. Quindi, credo che sia evidente facilmente comprensibile come le condizioni lavorative siano complicate. In merito vi è un'indagine della magistratura; abbiamo messo a disposizione tutti gli elementi in nostro possesso. Riguardo invece al grave evento che ha colpito l'area del Gargano nella giornata di ieri, e precisamente nei comuni di Vieste e Peschici, è opportuno fornire i più dettagliati elementi in merito, anche

la mobilitazione dei mezzi aerei) ha inoltrato al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile la richiesta di soccorso e su questo c'è stata una risposta una risposta immediata, in 40 minuti, attraverso l'elicottero Erickson S-64 con base a Pontecagnano, che ha raggiunto l'area di intervento alle ore 12,30, affiancato alle ore 11,58 da un altro S-64 di base a Pisticci. è arrivato il primo elicottero del nucleo di Bari dei Vigili del fuoco. Sul Gargano hanno operato, nel corso di tutto il pomeriggio del 24 luglio, tre elicotteri S-64, un elicottero AB-212 della Marina militare e due elicotteri CH-47 dell'Esercito, più due elicotteri dei Vigili del fuoco, facendo oltre 200 lanci di liquido estinguente. Sono stati utilizzati gli elicotteri in quanto, per queste particolari specificità (il Dipartimento di protezione civile così ha ritenuto dal punto di vista tecnico), era più utile utilizzare gli elicotteri Erickson, di grandi dimensioni e con una tipologia di lancio più precisa, piuttosto che i Canadair, che comunque erano impegnati in altre situazioni. A causa degli incendi in atto, va ricordato che la strada statale n. 89 è stata chiusa nel tratto costiero da Vieste a Mattinata, determinando gravi difficoltà nei collegamenti e anche nei soccorsi, così come l'autostrada Bari-Napoli; la strada statale che consentiva una viabilità alternativa è stata chiusa per una frana che ha coinvolto anche un camion cisterna che trasportava liquidi pericolosi. La popolazione evacuata è stata di circa 3.000 persone; ci sono stati numerosi interventi di solidarietà,

Carabinieri. L'evacuazione delle 3.000 persone si è svolta, comunque, in una situazione di grande collaborazione e di grande disponibilità. Le 3.000 persone, quelle di Scandicci più tutti coloro che da Vieste hanno trovato una sistemazione, sono state sistemate presso gli alberghi di San Giovanni Rotondo (1.339 persone, che sono state trasferite in pullman) negli alberghi dei Comuni di Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Mattinata, in cui risiedono rispettivamente 158, 151 e 190 persone che si sono mosse autonomamente utilizzando le loro autovetture. Una porzione consistente della popolazione ha invece deciso di non allontanarsi da Vieste (1.600 persone) e da Peschici (100 persone). Complessivamente, la popolazione evacuata è stata di 3.538 persone. C'è stato un grande lavoro anche di ricongiungimento dei nuclei familiari, che, come facilmente si può immaginare, era necessario dopo la fuga dalle spiagge. La situazione ha assunto carattere di notevole drammaticità quando, alle ore 16,50, è arrivata anche la notizia dei due morti carbonizzati in località Calo Lungo, lungo la litoranea Peschici-Vieste. Il Presidente del Consiglio ha naturalmente ritenuto indispensabile, con un proprio decreto, dichiarare l'eccezionale rischio di compromissione e quindi ha dichiarato lo stato di emergenza. del personale impegnato nell'emergenza di Foggia è stato di oltre 400 uomini tra l'Arma dei carabinieri, i Vigili del fuoco, le Forze armate e le Capitanerie di porto;

una quota infatti è arrivata anche dalle altre Regioni italiane, grazie allo spirito di solidarietà che caratterizza il nostro Paese. Anche la Regione Calabria è stata interessata dal fenomeno molto grave degli incendi boschivi e in questo caso la situazione è ancora abbastanza complicata. In questa Regione già nella nottata tra il 20 e il 21 luglio il fenomeno ha assunto particolare gravità.

ed urgente: questa mattina, infatti, 100 Vigili del fuoco che stanno completando il loro periodo di formazione (e hanno tutti i requisiti per poter intervenire) sono stati trasferiti urgentemente in Calabria.

Ci sono stati momenti di grande difficoltà in Provincia di Pescara e nelle zone di Scafa (Capoluogo) e di Bussi Officine. C'è stata un'interruzione della ferrovia, si sono avuti momenti difficili, in particolare nelle vicinanze delle industrie produttive della zona, dove la Solvay, un'azienda ad alto contenuto

Nella Provincia di L'Aquila, in particolare nell'area ricadente nell'altopiano di Navelli e Collepietro, ci sono stati eventi complessi che hanno visto impegnate tutte le forze della Forestale

nella notte tra il 23 e il 24, e nella giornata di ieri, si è sollevato un forte vento: l'indisponibilità di mezzi aerei nelle prime ore di intervento ha prodotto una situazione particolarmente complicata. I diversi comandi dei Vigili del fuoco e della Guardia forestale hanno lavorato in maniera coordinata, anche se nella Provincia di Nuoro si è prodotta una situazione

all'Azienda sanitaria di monitorare continuamente la situazione atmosferica ed abbiamo registrato concentrazioni significative di prodotti inquinanti.

anche qui c'è una forte competenza delle Regioni; competenza che va esplicata nel monitoraggio del territorio, perché un piccolo incendio avvistato rapidamente

bisogna aumentare il livello di prevenzione, così come alcune Regioni, in maniera assolutamente premiante, hanno fatto in questi anni.

gli strumenti a disposizione della magistratura prevedendo pene severe, come è importante mettere a disposizione migliori strumenti di indagine. Un altro elemento è costituito dalle forze dislocate sul territorio. Oggi non disponiamo di risorse sufficienti. Le nostre risorse sono sottodimensionate rispetto a questo tipo di emergenze. Sul territorio i Vigili del fuoco, ma anche la Guardia forestale, non hanno sufficienti mezzi e uomini per rispondere a questo tipo di emergenze. È bene saperlo, perché quando le emergenze sono contingentate e collocate in aree delimitate si possono far affluire uomini e mezzi dai comandi vicini; quando, invece, le emergenze sono così diffuse su tutto il territorio nazionale, questa operazione diventa molto più complicata. Abbiamo bisogno

devono essere risorse che coinvolgano il volontariato, un volontariato che abbia capacità, formazione e catene di comando chiare. Inoltre, dobbiamo essere dobbiamo essere sempre prudenti. Oggi posso dire che la situazione è sicuramente migliorata rispetto a quella di ieri. Abbiamo ancora alcune criticità in Sicilia, regione colpita fortemente nella giornata di ieri, in particolare nell'area del Messinese. Abbiamo però

sufficiente un piccolo cambiamento climatico, un piccolo mutamento del vento. Questo ci fa dire che la situazione oggi è sicuramente sotto controllo. Abbiamo i dispositivi presenti su tutto il territorio, ma c'è da parte nostra grande attenzione

esposto un quadro abbastanza esaustivo di una situazione, che naturalmente non fa piacere al Governo dover riportare. Rispetto a questi eventi, credo vi sia la necessità che tutte le istituzioni e la politica sappiano dare risposte coerenti. Siamo qui a disposizione per quanto il Senato vorrà indicarci.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova situazione di emergenza incendi rischia davvero di mettere in ginocchio la nostra penisola. Mi preoccupa molto questo "flagello fuoco" che, con proporzioni finora mai riscontrate, sta seminando terrore e morte in tutto il territorio, specialmente al Sud. Dell'ultima ora gli annunci sul Gargano, appena di ieri le notizie di Peschici, dove un intero pezzo di popolo ha affrontato il mare sfidando la sorte e nuvoloni tossici per tentare la via della fuga. Come al solito, non è mancato lo straparlare e tante sono le polemiche e i battibecchi tra le opposte forze politiche, la protezione civile e quanti non sanno giustificare il perché dell'inferno di fuoco. Non hanno fatto a meno di colpirsi - è il caso di dire - con fuochi incrociati di accuse, cercando di addossare colpe alle esigue postazioni fisse di soccorso e ai mezzi stanziali della Protezione civile, alla leggerezza dei sindaci circa l'assenza del catasto delle aree incendiate. I sindaci contro i ministri, ministri contro le alte autorità civili, la protezione civile contro i politici: mi domando, *cui prodest*? Non è il caso di accusare, è la volta di risolvere. Almeno in queste occasioni di assoluta emergenza bisogna bandire le ciance ed agire per refrigerare - non a caso uso questo termine - i cittadini coinvolti in tali tragedie. A loro tutto il mio cordoglio, la solidarietà, ma anche la garanzia di intervenire concretamente. In queste ore necessita una risposta immediata e una collaborazione fattiva da parte di tutte le istituzioni. Il rischio della vita accresce il concreto pericolo che, insieme al patrimonio boschivo, vada in fumo l'intera economia turistica del Paese, come ammoniscono i vertici dirigenziali della piccola e media impresa pugliesi, i quali devono essere sostenuti e coadiuvati È tempo che il Governo intervenga, considerato che tutte le indagini e le inchieste sono giunte a risultati aberranti, lasciando intendere ad azioni mirate, preparate e premeditate non già di poveri piromani, ma di criminali incalliti. Senza smettere di cercare i criminali, è fondamentale approntare una politica di maggiore prevenzione e contemporaneamente di inasprimento delle pene esistenti per i reati in questione. Non bastano i divieti di costruire sui terreni percorsi dagli incendi, né sono sufficienti gli sforzi del Corpo forestale che controlla e perlustra le zone a rischio; neanche fungono da deterrente ordini di sequestro, perquisizioni o arresti. Appropriata, dunque, l'informativa del Governo, chiamato a riferire sui malsani gesti dai quali si evince massima mancanza di senso civico, del bene comune, dell'ambiente come risorsa irrinunciabile. Auspico, pertanto, interventi molto più incisivi per fare in modo che la legge sia rispettata completamente, che le forze impiegate vengano potenziate e infine che, superata l'emergenza, si dia il via ad un tavolo tecnico che metta d'accordo enti, amministrazioni e istituzioni e affronti la situazione per risolverla una volta per tutte, senza aspettare l'inevitabile riproporsi della tragedia. PRESIDENTE.

certo il futuro non sarà migliore del presente. Quando si va a valutare la situazione dal punto di vista degli equilibri biologici e si dice che ogni anno l'estate è più calda

Per i rifiuti la mia idea era ancor più drastica con riferimento ai commissariamenti, non certo per i singoli funzionari, Certo, se una Regione non fa il suo dovere dovrà pur esserci qualcuno che interviene.

invece di comprare 131 F-35 a 40 milioni di euro l'uno per portare le bombe atomiche e fare la guerra

seriamente impegnati in un'azione di spegnimento degli incendi nel Sud del nostro Paese. Si tratta dell'ennesima emergenza: l'Italia è nuovamente a fuoco. È una situazione che purtroppo si ripete ogni anno e regolarmente ogni anno tornano le stesse polemiche sui ritardi, sul mancato coordinamento di chi deve intervenire, sulle competenze delle Regioni, dei Comuni e così via.

i Forestali regionali, i Vigili del fuoco e l'Esercito. Si deve verificare se negli ultimi interventi vi sono state delle responsabilità; se si sono verificati problemi di coordinamento; è bene che si sappia per poterli evitare in futuro.

Nell'emergenza degli ultimi giorni si è fatto ricorso anche agli uomini e ai mezzi dell'Esercito: si tratta di un fatto eccezionale, che dovrà essere meglio precisato ed inserito nelle norme sul coordinamento con le Regioni. Data la situazione che si ripete annualmente, al di là degli strumenti della prevenzione, sarebbe opportuno ampliare il parco dei mezzi a disposizione della Protezione civile. La legge n. 353 del 2000, richiamata poc'anzi, affida anche alle Regioni, anzi soprattutto alle Regioni, compiti fondamentali contro gli incendi boschivi e prevede la possibilità che anch'esse si dotino di flotte regionali di elicotteri, che, però, devono trovare finanziamenti attraverso il bilancio dello Stato, con il supporto decisivo, come competenza tecnica, del Dipartimento della protezione civile. A questo vorremmo arrivare quanto prima.

il sistema di sorveglianza del territorio risulta insufficiente. Non ci sono mezzi adeguati e uomini schierati sul territorio, a parte i forestali, che intervengono solo a cose fatte per la riforestazione. Le cause di queste situazioni che si ripetono costantemente sono prevalentemente da ricercare o tra chi agisce per la speculazione, o nell'organizzazione del lavoro precario nei boschi. Per i primi, per gli speculatori, vi è un disegno strategico e doloso chiarissimo, individuato anche dalla citata legge del 2000: gli speculatori fanno affari sui terreni bruciati, che poi possono edificare. Qui si deve accelerare - è una richiesta precisa - un intervento diretto del Governo sulle amministrazioni comunali perché applichino immediatamente la legge n. 353 del 2000, che impedisce di costruire sulle aree bruciate. Si badi bene - ed è giusto che il Governo rifletta su questo - che solo il 6 per cento dei Comuni ha dato vita al catasto degli incendi, che sicuramente porrebbe fine una volta per tutte agli scempi estivi. Per combattere i piromani non servono nuove leggi; basta applicare quelle che ci sono, visto che la citata legge del 2000 per la prima volta ha introdotto il concetto del reato autonomo e punito, nell'articolo 423-*bis* del codice penale, con la reclusione da quattro a dieci anni. La legge c'è, ma non basta. Ci vuole una corretta gestione del territorio:

Adesso si stanno premiando gli interventi, spesso costosi, per spengere gli incendi, mentre la scelta corretta è quella seguita da alcuni Comuni della Sardegna e della Calabria, in Aspromonte, dove la vigilanza delle aree boschive è stata affidata ad associazioni di volontariato e a cooperative di giovani che aumentano così il lavoro stabile contro il precariato nella tutela dei boschi e hanno interesse ad evitare che il bosco bruci, sulla base del meccanismo per cui i Comuni pagano per intero quanto stabilito dalle convenzioni solo nel caso che il bosco non bruci e detraggono da lì una somma per ogni incendio che si verifica. In sostanza, si deve puntare alla prevenzione e, invece di finanziare la riforestazione, che è stato il vero male di questi anni, si deve incoraggiare la vigilanza. Questo è un modo virtuoso che il Governo dovrebbe far proprio ed estendere a tutto il Paese. Questo è l'impegno con cui cercheremo di dare il nostro contributo per finanziare con la legge finanziaria questi progetti.

dieci persone ogni chilometro quadrato! Forse non vi rendete conto di cosa vuol dire. Se queste effettivamente facessero il lavoro di cui ho parlato prima, sarebbe assolutamente impossibile il

delle forze, mi permetto di far notare che uno Stato che ha 500.000 uomini in divisa, su 59 milioni di abitanti, e che in alcune Regioni ha 50.000-60.000 unità tra guardie forestali e operai forestali, non può definirsi sottodimensionato. Piuttosto, preferisce spendere i soldi in stipendi,

Signor Presidente, anche l'UDC si associa al dolore per le vittime, un dolore che forse potevamo evitare. Caro Sottosegretario, la situazione è drammatica, i numeri lo dimostrano. Siamo di fronte ad un'altra emergenza: ormai sono un po' troppe, in questo Paese. Lei ha fatto una relazione puntuale,

qui il collega Sodano) è stato sollevato tante volte, forse più da voi che da noi, ma i fatti poi dimostrano che queste restano vuote parole. Parliamo di prevenzione tecnologica: leggo da alcune agenzie

Si dice che mancano risorse: è vero, lo stiamo sostenendo, lo ha detto la collega De Petris e lo sottolineo anch'io. Mancano fondi per fare attività preventiva e colgo l'occasione per dire grazie a tutti i volontari a tutti i volontari che si sono attivati e si attivano da tanto tempo e magari molte volte non ce ne accorgiamo. Grazie al Corpo forestale che sta aspettando, come le forze dell'ordine, il carburante per far funzionare i propri mezzi, e l'espletamento di alcuni concorsi. A questo proposito voglio fare un inciso: dico grazie a tutte le persone che si comportano e lavorano seriamente, perché ovviamente ci sono anche quelli che, magari per mantenersi il lavoro, appiccano gli incendi, ma questo è un altro capitolo. Questa è una vicenda emergenziale che ha tanti risvolti: quello umano, perché abbiamo visto le vittime e gli evacuati;

poi il problema della criminalità, di cui qui si è parlato giustamente, e mi associo anche a tanti colleghi della sinistra che hanno detto che le leggi ci sono e vanno rispettate. Questo è il problema del nostro Paese: le leggi ci sono, ma spesso non c'è la capacità,

caro Governo, dietro alle Regioni, che hanno sicuramente grandi colpe: sono contrario alla frammentazione proprio perché rischia di ingenerare la possibilità di scaricare le colpe su altri. Quando parliamo di risorse, scusate la battuta, molte volte mi sembra di essere in uno di quei Comuni che quando preparano il piano neve mettono nel relativo capitolo risorse che poi non ci saranno, sperando che non nevichi. Purtroppo, ci stiamo accorgendo che gli incendi ci sono, sono sempre più numerosi e purtroppo gli interessi economici in questo tipo di attività criminale sono così rilevanti che non possiamo pensare che possa diminuire senza un intervento deciso e convinto da parte di chi governa. Non mi ripeterò su quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, ma il Governo dovrebbe domandarsi come mai da quest'Aula vengano tante perplessità da tutte le forze politiche, nessuna esclusa. tante perplessità che deve farsi un esame di coscienza e deve intervenire il più rapidamente possibile, perché qui non è che c'è da condividere o meno le conclusioni del Governo: queste queste conclusioni mancano, caro Sottosegretario. Cerchiamo di essere realisti: il Governo deve avere il coraggio e anche la capacità di intervenire con durezza, e non certo la capacità che abbiamo dimostrato nell'emergenza rifiuti in Campania o quella capacità che ci porta all'abbandono del verde nell'ottica della tutela del verde. Ha ragione il collega Galli: il verde va tutelato e difeso,

settori e argomenti, anche l'anno prossimo, quando l'emergenza sarà già scoppiata e non si potrà fare più niente, ci troveremo qui a chiacchierare e a non risolvere il problema. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e in particolare a nome della senatrice Maria Celeste Nardini, momentaneamente indisponibile vocalmente, e che teneva a fare questo intervento. Cercherò di farlo anche a nome suo. Un ringraziamento va al sottosegretario Rosato per la completezza anche del quadro che ha rappresentato all'Assemblea del Senato sulla gravissima situazione degli incendi nel nostro Paese. Voglio innanzitutto esprimere, a nome del Gruppo, il cordoglio alle famiglie delle vittime e dei feriti e un ringraziamento agli uomini impegnati in queste ore, anche in questo momento, mentre siamo qui a discutere al Senato, per spegnere ancora i focolai di incendi in giro per il nostro Paese, in particolare nel Sud Italia; nonché un ringraziamento ai tanti volontari che sono stati impegnati, anche ieri, come nel caso tragico di Peschici, in cui i volontari pescatori hanno dato una mano per mettere in salvo i turisti e i cittadini presenti in quel luogo. Ho molto apprezzato l'introduzione del Sottosegretario rispetto al binomio emergenza climatica-emergenza criminale. Credo che dobbiamo ragionare in questi termini e dobbiamo farlo sempre di più nei prossimi anni. L'emergenza criminale legata agli incendi è una pagina nera per il nostro Paese, che si ripete da vent'anni. Negli ultimi vent'anni è stato distrutto nel nostro Paese 1.100.000 ettari di superficie boscata: un'estensione superiore a quella dell'Abruzzo, per dare un senso anche della dimensione della gravità del fenomeno. Ma all'emergenza del fenomeno. Ma all'emergenza criminale legata agli incendi si aggiunge quella climatica. Dobbiamo sempre di più fare i conti con i cambiamenti climatici e con un'aridità delle nostre terre che, purtroppo, è un processo di desertificazione che avanza e che riguarda non solo il Sud d'Italia, ma che si estende fino al Centro e che nei prossimi anni, se non si interviene con misure di adattamento, sarà sempre più drammatico. Questo è un tema su cui riflettere anche rispetto alle misure da mettere in campo. evidente - lo dicevano colleghi quali la senatrice De Petris ed il senatore Bellini - che vi sono leggi dal 2000 nel nostro Paese che vanno nella direzione di colpire di colpire appunto le mani criminali. Gli incendi sono dolosi, non sono colposi. Ormai alla leggenda che il mozzicone di sigaretta incendia i boschi non ci credono più neanche i bambini: gli incendi sono per l'80 per cento dolosi, sono per mano criminale, e bisogna intervenire con più durezza anche facendo in modo che chi commette un reato sia poi individuato e consegnato alle Forze dell'ordine. Purtroppo questo non avviene perché c'è una scarsa collaborazione e i fenomeni avvengono spesso, in alcune aree del Paese, con la complicità delle grandi organizzazioni criminali che sono interessate ai lavori, agli appalti, soprattutto per il rimboschimento, ma anche per per poter spegnere gli incendi e per le speculazioni edilizie. Allora, bisogna fare di più rispetto alla legge che prevede l'impossibilità della costruzione per dieci anni. Ma per fare questo, come veniva già detto, c'è bisogno che i Comuni facciano il catasto delle aree incendiate. delle aree incendiate. Questo non è stato fatto fino ad oggi: solo il 20 per cento viene denunciato; l'80 per cento non viene sottoposto al catasto, per cui sono aree teoricamente soggette a possibili iniziative, come varianti al piano regolatore, per intervenire ancora lì, per favorire la speculazione edilizia. È evidente che questo è un tema rilevante. Ma credo che, a fianco a questo (ha ragione il collega della Lega), c'è bisogno di maggiore prevenzione, ma la prevenzione non è negata da una coscienza ambientalista di questo Paese; non è legata da politiche verdi, ambientaliste di questo Paese; anzi, è l'esatto contrario, perché i veri ambientalisti non si oppongono a che si facciano opere di mitigazione, di prevenzione boschiva, non chiedono che non si facciano le strade frangifiamma, che non si facciano gli interventi di pulizia del bosco e del sottobosco.

straordinario per il nostro Paese, concerne anche la possibilità di avere maggiori forze, soprattutto di Vigili del fuoco. Vi è una carenza di organico, ormai riconosciuta dallo stesso Governo. Si parla di 15.000 uomini; 3.000 uomini del Corpo forestale dello Stato; Regioni intere che lamentano l'impossibilità anche di avere risorse per pagare il carburante dei mezzi militari o per pagare gli affitti per le caserme dei Vigili del fuoco. E questo riguarda tutte le Regioni, dall'Umbria alla Calabria, alla Campania, alla Puglia, riguarda il nostro Paese. Bisogna fare di più e meglio. Questo chiediamo al Governo. Così come abbiamo apprezzato la prontezza con cui il Governo è venuto qui e ci ha riferito in modo compiuto su ciò che è avvenuto in queste ore, ci aspettiamo che nei prossimi mesi, quando discuteremo di finanziaria, ci sarà un atteggiamento diverso appunto in materia di emergenza ambientale ed emergenza criminale. Questo è l'impegno che chiediamo al Governo.

ai familiari di chi ha perso la vita e la gratitudine, come già ricordato da altri colleghi, ai Vigili del fuoco, al personale volontario, al personale della Protezione civile, delle forze di polizia e delle Forze armate impegnate nell'opera di soccorso. È però difficile, Presidente, parlare di disastro ambientale imprevisto e imprevedibile, come se ci fosse stata un'improvvisa grandinata. Credo sia auspicio comune di quest'Aula che i colpevoli materiali del rogo siano individuati e condannati, ma, al di là della rassegna stampa del Viminale, oggetto dell'informativa del Governo, le prime informazioni ci fanno ritenere, anche per quello che dirò tra un attimo, che possano esistere responsabilità non soltanto da parte dei piromani, ma anche istituzionali, le quali esigono non che ci si divida ma che si ponga riparo nel più breve tempo possibile. Il Sottosegretario di Stato ricordava la legge n. 353 del 2000, che assegna alle Regioni e ai Comuni la competenza per la lotta agli incendi boschivi. In base a questa legge, se c'è un incendio non interviene immediatamente la Protezione civile: le segnalazioni vengono fatte pervenire alla sala operativa della Regione, che può chiedere l'intervento della flotta aerea dello Stato. Il dottor Bertolaso, persona seria e stimata da tutti, fuorché dal Governo in carica, che lo ha costretto alle dimissioni in Campania, aggiunge, da responsabile della Protezione civile, che nel giugno di quest'anno - lo ricordava anche il Sottosegretario - ci sono state due direttive del Presidente del Consiglio rivolte a Regioni, prefetture e Ministeri competenti, contenenti l'esortazione a far funzionare le sale operative delle Regioni per garantire un efficace coordinamento. venerdì 20 luglio, lo stesso dottor Bertolaso ha segnalato ai medesimi enti l'ondata di caldo che sarebbe arrivata, sollecitando l'adozione di piani di emergenza. Leggo sul «Corriere del Mezzogiorno» di oggi: «In Puglia, in autunno, sarà creata una struttura di Protezione civile sul modello di quella nazionale, in grado di gestire una rete di volontariato organizzata e coordinata». Sono parole riportate tra virgolette pronunciate ieri dal presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Lo stesso Vendola, in data 10 novembre 2005, quasi due anni fa, aveva dichiarato: «Entro pochi mesi anche la Puglia avrà un struttura regionale di protezione civile per prevenire e monitorare gli eventi calamitosi e formare la rete del volontariato». Sono passati molto più di pochi mesi: perché non è stato fatto nulla? La risposta a questa domanda va data in varie sedi. Dovrà essere data davanti all'autorità giudiziaria, se è vero che la procura della Repubblica di Lucera ha aperto un'indagine, non soltanto sugli eventuali piromani ma anche - cito testualmente - sui "tempi di arrivo e l'impiego dei soccorsi". andrà data in modo esaustivo anche in Parlamento. E perché non si dica che è facile parlare con il senno di poi, Presidente, vorrei ricordare che insieme al presidente Matteoli il 19 dicembre dello scorso anno, parliamo di sette mesi fa una lunga e articolata interrogazione sul Parco del Gargano, denunciando in quella circostanza la presenza soltanto di 40 agenti del Corpo forestale dello Stato, inclusi il comandante e il personale amministrativo, per un'area vastissima, non solo per estensione ma anche per numero di abitanti: 121.000 ettari e 210.000 abitanti. Denunciavamo il bilancio inadeguato e la carenza di personale. Purtroppo, non solo non è stata data risposta a questa interrogazione, ma non la si è data neanche nei fatti. Signor Presidente, noi non vogliamo avere ragione sette mesi dopo, esigiamo però risorse pubbliche adeguate e investimenti per la sicurezza. È inutile fare auspici, colleghi, per la prossima legge finanziaria: tra qualche minuto inizierà la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, nel quale non c'è una parola concreta sui temi della sicurezza e della prevenzione: tutto il resto è soltanto retorica!

un pensiero affettuoso per i morti e per i feriti e un pensiero di gratitudine per i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Forze armate, la Polizia e i Carabinieri, che si sono spesi non poco per questi eventi eccezionalissimi. Ma perché sono così eccezionali, questi eventi? Noi che ricordiamo quanto costò all'Italia la forestazione e sappiamo quanto fu virtuoso quel progetto di forestazione (si pensi per un momento agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nelle contrade dell'Avellinese, dell'Avellinese, agli interventi sull'arco alpino e sull'Appennino), ricordiamo che allora non c'erano incendi di queste dimensioni e pur tuttavia si costruiva il parco forestale italiano, che è diventato ricchezza e ha prodotto reddito ed occupazione. Ma evidentemente quella era una stagione nella quale i Governi riservavano al tema più attenzione di quanto non accada oggi: c'era attenzione non soltanto per la forestazione (vale a dire per l'impianto), ma anche per la manutenzione, la custodia, l'acquisizione delle risorse idriche necessarie per svolgere l'indispensabile prevenzione, l'attività necessaria per consentire, per quanto possibile, la fruizione dei boschi e delle foreste italiane. I danni che si sono verificati in questi giorni, rappresentante del Governo, non hanno precedenti e, così come ha detto qualcuno prima di me, anche le Regioni, e più segnatamente la Regione maggiormente danneggiata, la Puglia, avrebbero potuto e dovuto adottare preliminarmente i provvedimenti del caso. In queste ore e in questi giorni ci occuperemo della finanziaria, ma ci occuperemo anche del cosiddetto tesoretto. Non scordatevi che ciò che si incendia solitamente è il patrimonio boschivo demaniale, quello dei privati non si incendia; se ciò non accade è perché colà c'è una manutenzione che nel patrimonio pubblico non esiste. Occorre quindi fare la manutenzione, laddove c'è l'erba, laddove c'è il sottobosco, ci può essere l'incendio; nelle proprietà private gli incendi non si verificano così facilmente. E allora attenzione: finanziamenti subito, se non si vuole che l'anno prossimo si ripetano eventi come quelli che sono accaduti.

strutture necessarie per la manutenzione, per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile, e chiunque ha responsabilità sappia che non può piangere sul latte versato come sta accadendo in Puglia.

per qualche chiarimento in merito all'interrogazione che avevo presentato. In primo luogo, esprimo il sentimento di cordoglio alle famiglie delle vittime, che poi non sono due, purtroppo, perché ce n'é una terza, non a Peschici o Vieste, ma da un incendio non ricordato dal Sottosegretario, quello di Rocchetta Sant'Antonio: si tratta del morto che si è registrato sull'autostrada a causa degli effetti dell'incendio stesso. stesso. Nell'interrogazione orale chiedevo qualche chiarimento per ciò che attiene alla dinamica degli interventi e ai tempi degli interventi stessi.

perché si ipotizzano ritardi eccessivi anche in un contesto, quale quello del Paese intero, sottoposto ad uno *stress* molto forte da questo punto di vista.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, è mia volontà esprimere il plauso alla Protezione civile e a tutte le istituzioni per la qualità dell'intervento, ieri, nel territorio di Peschici e del Gargano e delle altre Province italiane. Data la mia provenienza, colleghi, mi perdonerete, mi soffermerò soprattutto sul Gargano. Le cronache anche questa mattina (bastino per tutti i servizi del TG1 delle ore 13,30) testimoniano, attraverso le voci di chi era sul luogo del disastro e dei rappresentanti locali, che i soccorsi ci sono stati e sono serviti per garantire l'assistenza necessaria *in primis* alle persone. Detto questo, chiarezza sui tempi circa tutto l'evolversi della tragedia, dalle prime segnalazioni ufficiose a quelle ufficiali, dev'essere fatta con ogni solerzia, per capire se vi siano responsabilità. Oggi, la terra di Capitanata piange una delle sue tragedie più grandi. Seppure i danni alle persone (voglio rinnovare il mio cordoglio e quello di tutti i senatori dell'Ulivo alla famiglia delle due vittime di ieri) non hanno avuto dimensioni da cataclisma, ciò che è accaduto rappresenta una ferita lacerante: economica, sociale e soprattutto morale, per tutti gli abitanti della Provincia di Foggia e del Gargano in particolare. Credo che gli eventi drammatici di ieri abbiano riportato alla memoria di tanti foggiani le immagini della tragedia di viale Giotto del 9 novembre 1999. Ieri è stato distrutto (e bisognerà assolutamente accertare se in questo c'è stato dolo o qualche disegno criminale, come sempre accade nel caso degli incendi in Italia) un pezzo della terra di Capitanata, il territorio più rappresentativo della Provincia. I danni alle infrastrutture, al comparto turistico, all'agricoltura e al patrimonio ambientale sono immani. Ecco perché ritengo necessario un intervento immediato del Governo per formalizzare lo stato di calamità naturale e garantire così la ricostruzione. Insieme a tale riconoscimento, è indispensabile lo stanziamento di risorse urgenti per evitare che la stagione estiva venga compromessa del tutto, con la drammatica conseguenza di infliggere un colpo mortale alla stessa sussistenza di centinaia di famiglie. Assume urgenza immediata ed improcrastinabile la previsione di interventi fiscali, previdenziali e bancari che possano assicurare alle famiglie e alle imprese la possibilità di ricostruire i loro beni distrutti dai roghi. Le immagini e le testimonianze sulla tragedia di ieri, gentili colleghi, dove è emersa la necessità di rafforzare i presìdi di prevenzione con una presenza maggiore di infrastrutture, mezzi e uomini, in particolare dei Vigili del fuoco (ringrazio il dottor Rosato, che ieri si trovava nella Provincia di Foggia, dove ha sottolineato la carenza di queste strutture), impongono un impegno immediato anche per la fase di ricostruzione, che dev'essere tempestiva, concreta e soprattutto efficace, per evitare qualunque forma di speculazione. Ecco perché è mio convincimento e di tutti i colleghi dell'Ulivo, visto anche il brillante ed operativo lavoro svolto ieri dall'unità di crisi costituita alla prefettura di Foggia, sotto la direzione del prefetto Sandro Calvosa (che ringrazio), il quale ha assicurato il coordinamento e la diffusione delle notizie sulla tragedia, che debba essere immediatamente formalizzato un coordinamento territoriale e provinciale che gestisca la fase di ricostruzione. Il territorio colpito dal fuoco, gentili colleghi, e bruciato sotto gli occhi dell'intera Nazione è un territorio complesso, dove insistono diverse istituzioni: Comuni, Provincia, Regione, Comunità montana e Parco del Gargano. E appaiono molto strumentali le parole del presidente del Parco del Gargano che, fuori dal coro, scarica sugli altri le responsabilità della manutenzione del Parco. Deve essere Deve essere altresì impegno del Governo evitare ciò che è accaduto in altre sciagurate circostanze, dove all'emergenza e alla ricostruzione si è risposto con la deriva delle responsabilità. La gestione e il coordinamento degli interventi di ricostruzione deve essere assicurato dalle istituzioni provinciali che, avendo una visione autentica e d'insieme delle esigenze e delle priorità, possa garantire efficaci azioni di sostegno alle popolazioni colpite. Ritengo, colleghi tutti, che su questo non ci possano non essere ampie convergenze.

non risulta che il Governo abbia presentato nell'ambito del DPEF - ed è un obbligo di legge programmatica relativa alle entrate e alle spese delle pubbliche amministrazioni, cioè il dato fondamentale di riferimento dell'intera architettura di politica economica. Senza tali tabelle, francamente, non capisco in che modo si possa svolgere il dibattito, né di cosa discutiamo.

È evidente che se si scrive che l'obiettivo per il 2008 è un *deficit* del 2,2 per cento, bisogna sapere se quell'obiettivo è perseguito come proposta del Governo - aumentando la spesa e aumentando le entrate o riducendo la spesa e riducendo le entrate. Se non c'è questo dato, ritengo che la discussione generale sul DPEF sia assolutamente priva di senso. Lo avevo già detto in Commissione e ci era stato assicurato che in corso d'opera il Governo avrebbe provveduto, ma alle ore 17,30 di oggi questo dato non esiste, non è stato ancora presentato in Aula.

perché nel DPEF presentato al Parlamento è scritto con chiarezza che quei dati numerici scontano la presenza del cosiddetto scalone Maroni;

oltre alla mancanza delle tabelle di entrata e di spesa della pubblica amministrazione, senza le quali l'obiettivo dei saldi è ingiudicabile, c'è, come novità rispetto al momento in cui è stato presentato il documento, un elemento in più palesemente scritto nel DPEF. I numeri contengono lo scalone Maroni

Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta e farò alcune brevi integrazioni, riprendendo anche la discussione che si è svolta in Commissione, e tentando di offrire pure alcuni spunti di riflessione attorno alla risoluzione che poi alla fine approverà questo Documento di programmazione economico‑finanziaria. Penso che sia mio dovere fornire una valutazione circa la cosiddetta manovra lorda. Come avete visto dal documento, è una manovra che potrebbe ammontare a 21 miliardi di euro: in ogni caso, ribadisco subito che il Parlamento siamo noi e decideremo l'ammontare, cosa fare e cosa non fare, e soprattutto quali

operare attraverso la *spending review*, che può portare a risparmi significativi, e superare il concetto della spesa storica. Sotto questo versante ritengo, signor Presidente, che il Documento di programmazione economico-finanziaria di quest'anno una caratteristica rilevante, nel senso che è molto trasparente, sicuramente molto più trasparente dei precedenti Documenti, perché nel Documento in esame vengono indicate precisamente le spese che non sono previste dalla legislazione vigente. È il Parlamento, come dicevo prima, che deciderà e aumenta, in questo caso, la sua capacità, il suo dovere, il suo diritto di intervenire su tali questioni.

vi sono spese derivanti dalle prassi consolidate (per esempio i contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato, delle Poste) ed ipotesi, per così dire, relative a nuove iniziative. Per esempio, sappiamo che all'interno della maggioranza e del Governo da tempo si discute della necessità di intervenire riducendo l'ICI sulla casa ed anche da questo punto di vista è opportuno che si indichino in modo preciso le iniziative che devono essere finanziate. Credo che questa sia una novità assoluta: si finanziano le spese attraverso la qualificazione della spesa stessa, partendo dalla spesa primaria. Anche perché l'obiettivo, ribadito più volte, è di fermare l'aumento della pressione fiscale, anzi gradualmente di diminuirla. Quindi "no" a finanziamenti di spese attraverso l'aumento della pressione fiscale. Questo è un tema che è stato oggetto anche di discussione nella Commissione bilancio. Ribadisco che è impegno sia del Documento di programmazione economico‑finanziaria che della maggioranza di operare perché la pressione fiscale venga gradualmente diminuita nei prossimi anni. È una scelta, ritengo, indirizzata alla sostenibilità finanziaria e alla sostenibilità ambientale. Per le nuove iniziative ritengo un ruolo importante, rilevante debba assumere il Protocollo di Kyoto: lì c'è la riforma energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il risparmio, l'efficienza, un sistema più democratico perché basato sul consenso e sulle esigenze del territorio per l'individuazione dei siti e per la realizzazione delle opere. Poi l'uso della fiscalità per incentivare comportamenti virtuosi sul piano energetico e per penalizzare le fonti inquinanti. L'ambiente non è più solo un vincolo, l'ambiente diventa una grande opportunità per costruire un progetto di sviluppo, per costruire un'idea di sostenibilità che renda il nostro Paese più competitivo, in grado di vincere le sfide della competizione globale. poi la manovra sull'ICI. Mi auguro che nella risoluzione della maggioranza vi sia una indicazione in tal senso per venire incontro ai proprietari di casa in modo equo e sostenibile. Sappiamo che circa l'80 per cento dei cittadini italiani sono proprietari di casa, ovviamente non è qui il caso di entrare nel dettaglio, cioè sui criteri per realizzare questa manovra (per esempio, un tetto di reddito o la superficie

nei confronti dei ceti più poveri, bisogna intervenire a favore di chi deve pagare l'affitto. Questo credo debba essere un impegno che tutti dobbiamo assumerci. C'è inoltre la questione della tassazione

operazioni deve essere destinato nella stessa operazione a sostegno dei redditi più bassi, ad esempio per le famiglie che abbiano in casa anziani incapienti o non autosufficienti. Presidente, rispettiamo i parametri di Maastricht (il nostro Paese è rientrato entro i parametri di Maastricht); rispettiamo il piano di rientro che è stato adottato nella precedente legislatura; siamo nel 2007 al 2,5 per cento di *deficit* in rapporto al prodotto programmatica prevedeva il 2,8, quindi siamo ampiamente sotto), compreso il il costo del decreto extragettito che esamineremo la prossima settimana. Nel 2008 arriveremo al 2,2, senza manovra correttiva, perché il tendenziale è uguale al programmatico. Nel 2008 riteniamo si debba chiudere la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese - ripeto - adottata nella

è come se ci fosse una redistribuzione indiretta, dal momento appunto che non c'è l'esigenza di operare con una manovra correttiva. Si crea una situazione per la quale c'è più libertà da parte di tutti gli organi che attengono alla definizione di tali questioni e anche del Parlamento, c'è più libertà nella scelta delle politiche economiche, economiche, viene meno l'assillo del reperimento delle risorse per la manovra correttiva, perché c'è la stabilizzazione della finanza pubblica. In questo senso credo che il Parlamento abbia più responsabilità,

ora ha il Parlamento, sarebbe sbagliato sottrarsi, lo possiamo e lo dobbiamo fare se manteniamo fermi i vincoli di non aumentare le tasse e di qualificare, migliorare e rendere più produttiva la spesa primaria.

È stato anche posto il problema del perché rinviare agli ultimi anni, fino al 2011, il risanamento finanziario. la Commissione europea nei periodi di crescita economica occorre spingere di più sul risanamento, come mai in Italia avviene il contrario? Come mai si rinvia

perché i soldi maggiormente incassati, derivanti dalla crescita economica, sono tutti finalizzati alla riduzione del *deficit*

liberalizzare i mercati per creare effetti positivi sui prezzi e rendere il Paese e i mercati più competitivi, creare una sana

Non solo più *welfare*, ma anche più efficienza ed efficacia nella spesa. Ritengo che sia positivo l'accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali per la produttività

esame rinuncia completamente ad effettuare qualsiasi tipo di intervento perché deve in qualche modo lubrificare la pace sociale o meglio politica all'interno delle forze della maggioranza, deve concedere qualcosa ed avviare una politica di spesa facile che normalmente contraddistingue i periodi pre-elettorali.

seri quest'anno e l'anno prossimo, si rinuncia e si rinvia, con l'ovvio risultato che nel 2009 bisognerà fare un intervento di almeno dieci miliardi di euro; nel frattempo, però, si dà corso alla spesa.

dilazionare un po' il risanamento, facendo però contemporaneamente ripartire il Paese con un potente intervento di detassazione, sarebbe stato comprensibile; non è, però, comprensibile che si dilazioni il risanamento per allargare i cordoni della borsa. Francamente ciò significa peggiorare la situazione del Paese negli anni futuri.

veramente notevole di ridurre la spesa pubblica (è possibile, ma 20 miliardi di riduzione non sono bruscolini, quindi è molto difficile), se non altro, però, l'esperienza dovrebbe dimostrare che è difficilmente attuabile. Il Governo attuale si vanta di aver prodotto nella finanziaria per il 2007 un comma, il 509, nel quale erano previsti oltre 4 miliardi di tagli alla spesa dei Ministeri. Il risultato è che

della spesa pubblica, trascurando il piccolo particolare che non è con una revisione o un'operazione di abbellimento, di riconsiderazione che si riduce la spesa pubblica, ma la spesa pubblica si riduce intervenendo sulla legislazione sostanziale di spesa, su singole leggi e cancellando prestazioni ed interventi, uno per uno, non semplicemente facendo riferimento alle compatibilità dei singoli Ministeri. Tra l'altro, sappiamo tutti che ogni Ministero è geloso della propria spesa e non intende diminuirla.

A parte il fatto che la pressione fiscale è già aumentata di due punti nell'ultimo anno e mezzo e fa dell'Italia uno dei Paesi in cui le tasse sono più elevate rispetto al resto dei nostri concorrenti, questo significherà aumentarla ulteriormente e quindi pregiudicare ancora le possibilità di sviluppo. Nel DPEF si la pressione fiscale andrà gradualmente calando. A parte che la previsione di un calo di 0,2 punti nel corso del quinquennio è sostanzialmente risibile, dobbiamo porci il problema se,

da interventi, a mio sommesso avviso, alquanto punitivi: interventi retroattivi, che considerano redditi quelli che una volta erano costi di produzione per le imprese, interventi che concernono le famiglie e che colpiscono i ceti medi. Infatti, modificare la curva dell'aliquota IRPEF, iniziando a "mordere" intorno ai 30.000 euro netti, non significa colpire i ricchi; significa colpire non dico i poveri, ma chi è appena in grado di sopravvivere.

di parte governativa, come la lotta all'evasione, la redistribuzione e lo sviluppo sostenibile, sono forse astrattamente condivisibili da un punto di vista lessicale, ma in concreto mostrano

facendo pagare prima di diminuire la tassazione, ciò significa spremere molto di più e mandare molte imprese e molti contribuenti fuori mercato. Il recupero della lotta all'evasione, invece, ha senso - ed è stato fatto nel passato - abbassando le aliquote nominali, in modo da rendere anche meno conveniente e

Anche la favola della redistribuzione non funziona. Non è redistribuendo un reddito con il meccanismo dell'invidia sociale, signor Presidente, che si crea ricchezza. La redistribuzione può avere senso se c'è sviluppo; se non c'è sviluppo, c'è poco da redistribuire, c'è una lotta tra poveri che non porta ad un miglioramento complessivo del tenore di vita dei cittadini. Quanto allo sviluppo sostenibile, facciamo attenzione. Sicuramente dobbiamo adottare comportamenti compatibili con l'ambiente, però bisogna anche rendersi conto che adottare acriticamente alcuni parametri (mi riferisco principalmente al Protocollo di Kyoto) che penalizzano le nostre imprese proporzionalmente in modo maggiore rispetto a quelle dei Paesi nostri concorrenti determina costi che difficilmente possono essere sopportati dal nostro sistema di imprese. Quindi, facciamo attenzione agli *slogan* e valutiamo concretamente quello che sta attivandosi in questo Paese. Per completare il ragionamento sugli obiettivi di finanza pubblica, non si può non sottacere come questo Governo non indichi nessuna iniziativa per quanto concerne quanto concerne la riduzione dello *stock* del debito. Non c'è un'iniziativa relativamente al tema delle privatizzazioni; sui servizi pubblici locali si affida tutto ad un disegno di legge che torna sostanzialmente al passato; su interventi di diminuzione dello *stock* del debito, con qualche *swap* o strumenti di questo genere per ridurre genere per ridurre il costo degli interessi (tanto più che siamo in una fase di crescita dei tassi), nulla si accenna. Questo rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per il futuro.

La rimozione dello scalone, oltre a rinviare all'infinito l'aggiustamento del sistema pensionistico, è ottenuta con costi notevoli (quantificati in 10 miliardi, ma vedremo se saranno di più), sulle spalle di una redistribuzione della spesa pensionistica all'interno del settore, per esempio aumentando i contributi dei lavoratori parasubordinati. Ciò, in soldoni, vuol dire che consentiamo un miglior trattamento agli anziani penalizzando i giovani, il che da un punto di vista sociale generale mi sembra moralmente non condivisibile. Non era questo

alcune infrastrutture sono viste come una sorta di accordo politico. Il Governo ha ribadito la volontà di completare l'Alta velocità tra Torino e Lione, che però costerà un miliardo in più, semplicemente per - come dire - lubrificare il consenso. Mi domando se tutti i contribuenti trovino grande beneficio da questo tipo di accordo. La stessa considerazione riguarda il federalismo fiscale. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di passare ad un meccanismo di federalismo fiscale, però questo avrebbe senso nell'ambito dell'invarianza complessiva del gettito, perché in fondo è sempre il contribuente che paga per lo Stato, per la Regione, per la Provincia e per il Comune. Conferire a Regioni, Province e Comuni nuovi poteri di imposizione, e soprattutto la ricerca di nuove basi impositive, significa significa incentivare la crescita della tassazione e quindi gravare ulteriormente sugli stessi contribuenti (già colpiti da una serie di misure, non ultime quelle della scorsa finanziaria) e pregiudicare ancor di più le possibilità di sviluppo del Paese. In conclusione, signor Presidente, questo Documento di programmazione è privo di qualunque volontà di contrastare una realtà che si vede come crepuscolare e di declino. In sostanza, il Governo china la testa davanti ad una situazione di difficoltà (che nessuno si nasconde), anziché affrontarla.

di pace politica all'interno della variegata composizione della maggioranza, ci si arrende al declino, si accetta l'ineluttabile e si rinuncia a fare qualunque cosa. Per concludere, come ha detto il relatore di maggioranza, credo che si potrebbe anche arrivare ad una crescita del 3 per cento del PIL, che sarebbe un obiettivo

la mentalità di chi governa attualmente l'economia, di superare quei condizionamenti politici che portano a preferire una politica di redistribuzione e di pace politica, piuttosto che una politica aggressiva e di sviluppo. In sostanza,

Signor Presidente, colleghi, il Senato è chiamato oggi ad affrontare il primo appuntamento della manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011. Si pronuncerà, infatti, sul Documento di programmazione economico-finanziaria, utile base di confronto e discussione per il Parlamento sulle linee di politica economica e finanziaria del Governo. Un documento caratterizzato, come lo scorso anno, dall'efficace impostazione «sviluppo-equità-risanamento» e che prevede come presupposto la strategia dello «spendere «spendere meglio». Una strategia assolutamente condivisibile e che permetterà di recuperare risorse preziose all'interno del bilancio, a favore della qualità e dell'efficienza della spesa. Una strategia sulla quale il Parlamento ha già iniziato a lavorare, basti pensare alle recenti determinazioni sulla riduzione dei cosiddetti costi della politica. Come più volte ha sottolineato il ministro Padoa-Schioppa, non si è abbandonata la via del risanamento, infatti sono stati pienamente onorati e continueranno ad essere rispettati gli impegni sottoscritti in sede europea nel 2005. Questo però non significa che i problemi economico-finanziari del Paese siano finiti. Non a caso il Ministro, in un recente convegno, ha descritto l'Italia come «un'azienda fortemente indebitata e sottocapitalizzata», che paga anche i costi di una diffusa evasione fiscale che sottrae alle casse dello Stato circa 100 milioni di euro all'anno, influendo negativamente sulla redistribuzione del carico fiscale e alimentando gravissime distorsioni del mercato. Oggi, tuttavia, possiamo chiaramente affermare che l'emergenza dei conti è cessata. Ed è per questo che il Governo, rispondendo responsabilmente alle esigenze avvertite e chiaramente manifestate dai cittadini sfiduciati, ha inteso inserire nel DPEF

che i cittadini percepiscano concretamente i risultati che la politica economica di questo Governo ha raggiunto in poco più di un anno di lavoro; che si rappresenti la realtà economica italiana basandosi su dati e cifre certe, e non su interpretazioni facilmente strumentalizzabili; che si ricominci a dialogare con il Paese, recuperando la frattura che c'è stata con l'opinione pubblica. In questo senso, l'Udeur si è fatto più e più volte sostenitore con l'Esecutivo di alcune proposte che rappresentano le istanze delle famiglie italiane: le istanze delle famiglie che stentano ad arrivare alla fine del mese, secondo un dato allarmante che ha visto innalzarsi la soglia di indigenza; le istanze dei giovani che vorrebbero formare una propria famiglia, ma non riescono a causa della precarietà del lavoro e della difficoltà di trovare una casa. Recependo queste nostre proposte, il DPEF, nella parte relativa alle politiche per l'equità sociale, dedica un capitolo al piano nazionale per la famiglia che comprende proprio: il sostegno dei redditi dei nuclei meno abbienti; l'agevolazione all'accesso dei servizi per le famiglie più numerose, anche attraverso la revisione dell'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente); la conciliazione delle responsabilità familiari con il lavoro, tramite nuovi asili nido; un istituto per il sostegno del reddito alle famiglie con figli minori. Viene inoltre confermato l'impegno, a partire dal 2008, di ridurre l'ICI sulla prima casa - che auspichiamo possa trasformarsi presto in abbattimento totale - e di agevolare i giovani per l'acquisto o l'affitto dell'abitazione. Questi naturalmente sono solo alcuni dei contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria; alcuni degli impegni del Governo che la maggioranza parlamentare, approvando il suddetto documento, ribadisce nella risoluzione sulla quale preannunzio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Misto-Popolari-Udeur. Vorrei concludere il mio intervento, auspicando che la legge finanziaria per il prossimo anno traduca efficacemente le linee di intervento indicate nel al fine di gettare le basi per un'ulteriore crescita del Paese. *(Applausi dei Signor Presidente, onorevole sottosegretario Sartor, questo Documento di programmazione economico-finanziaria sottende ad una impostazione strategica quasi da "fine legislatura", in quanto appare di breve respiro, direi rinunciatario. Non a caso è stato oggetto di dure reprimende da parte di organismi internazionali e giudizi negativi da parte di istituzioni pubbliche come l'ISAE, la Banca d'Italia e la Corte dei conti. La presunta crisi dei conti del 2006 è servita solo a realizzare una manovra 2007 sbagliata, nei tempi e nei modi, per costruire quel fondo utile per il cosiddetto risarcimento sociale che avete propugnato. C'è una contraddizione evidente tra i richiami del ministro Padoa-Schioppa alla crisi della finanza pubblica, paragonata a quella del '92-'93, e le scelte che vengono operate oggi. C'è un parallelo evidente, invece, con l'errore storico compiuto nella fase '83-'87, allorquando il ciclo economico favorevole, condizionato dall'eccessivamente oneroso cambio lira-marco, determinò una crescita esponenziale del debito pubblico e non fu utilizzato a pieno per riforme strutturali, a parte la grande scelta sulla scala mobile e sulle indicizzazioni che hanno avuto benefici effetti sulla tenuta del sistema. Per le differenze profonde e la conseguente difesa degli egoismi della coalizione, oggi voi state compiendo lo stesso errore di allora. Viene pesantemente vulnerato il percorso di correzione dei conti pubblici, come ha rilevato anche il presidente Dini da cui ci aspettiamo una iniziativa coerente nella risoluzione, attraverso questo inutile DPEF, e conseguentemente delle riforme strutturali poiché rivede l'obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL; ammesso e non concesso che sia realistico anche al netto delle operazioni di *roll-over*, ormai una costante delle decisioni di bilancio. Contemporaneamente, il decreto-legge n. 81/2007 "affiancato" al DPEF, con una manovra di carattere espansivo, comporta un chiaro peggioramento del tendenziale e del *deficit* di 0,4 del PIL, azzerando i pochi risparmi prodotti dalla finanziaria 2007. Non vi rendete conto che l'Italia viaggia con un rimorchio attaccato e che occorre alleggerire il carico del debito pubblico, che impedisce una più forte velocità di crociera. Nello scenario di ripresa economica in atto, l'Italia si colloca su valori di crescita tendenziali decisamente più limitati, a conferma della strada ancora lunga da percorrere sulla via delle riforme di liberalizzazione dei mercati e di incentivazione della concorrenza.

determinando un livello insopportabile per la competitività delle imprese, per le famiglie e per i contribuenti. Evidentemente il Governo Prodi tiene moltissimo a questo ambizioso traguardo. E per i cittadini che pagano e continuano a pagare le tasse si arriva ad una pressione fiscale che supera il 52 per cento. È completamente assente nel dibattito la questione della pressione fiscale. La maggiore pressione identificata come strutturale sarà in un certo senso ipotecata per coprire interventi di aumento strutturale della spesa, in particolare di quella corrente. Avete vinto le elezioni con una serie infinita di promesse; ora continuate a ingannare gli italiani con promesse di minori tasse, di minore pressione fiscale, che non c'è, che non ci sarà, perché alimentate soltanto nuova spesa improduttiva. Comunque, dove nei Paesi più sviluppati si è ridotta l'evasione, lo si è fatto riducendo le aliquote e la base imponibile per rendere più conveniente pagare le tasse. Siamo preoccupati per la riforma del catasto, perché colpirete pesantemente il bene casa. I contribuenti saranno nell'impossibilità di impugnare le tariffe d'estimo e di verificare la loro congruità davanti ad un giudice terzo, affidando la decisione sulle rendite catastali ai Comuni. È come mettere una volpe in un pollaio. Risultano assenti le quantificazioni per i prossimi rinnovi contrattuali. Non avete alcuna intenzione di ridurre la spesa improduttiva e gli sperperi; non affrontate la competitività del sistema Italia. Risulta assente la questione previdenziale sia rispetto alla finestra di opportunità sia rispetto all'equilibrio previdenziale di lungo periodo (che tenga conto dell'andamento del tasso di natalità, delle aspettative di vita, del tasso di dipendenza degli anziani sopra i 65 anni, della crescita della spesa pubblica, del vincolo di bilancio) per i riflessi che hanno sulla sulla finanza pubblica e sulla spesa sociale. Non vengono fornite indicazioni, inoltre, né sulle eventuali risorse da destinare all'accordo sullo scalone, diventato scalino, né su quanto viene reperito nell'ambito del sistema previdenziale, né quanto recuperato nell'ambito delle cosiddette nuove iniziative. E l'accordo sugli scalini dimostra la fragilità dell'intesa, che non ha retto un giorno vista la pronuncia della CGIL, che non può che essere valutata negativamente e che comunque deve essere incorporata in questo DPEF, perché non c'è; non può essere demandato solo alla legge finanziaria, con un Parlamento espropriato con il ricorso ai voti di fiducia da parte di chi vuole imporre al Parlamento quell'accordo che si scarica sulla finanza pubblica, perché aumentano i costi e vi sono rischi sulla copertura. Aumentate le aliquote contributive e sulla razionalizzazione degli enti previdenziali siete talmente incerti sul risultato che avete inserito la clausola di salvaguardia, prevedendo ulteriori inasprimenti. inasprimenti. Questo accordo è più vicino a quello del 1975 che non a quello di San Valentino. Epifani oggi si sta defilando e Carniti ebbe certo più coraggio di quanto non ne abbia oggi Bonanni. Si seguita ad espropriare i lavoratori di diritti derivanti da norme come è avvenuto per il TFR, che, è bene ribadire, è salario differito. Mancano indicazioni sulle determinanti del maggiore gettito realizzato nel 2006, che costituisce la base revisionale per il 2007 e gli anni successivi, nonché i risultati dell'attività di contrasto all'evasione, atteso che la legge finanziaria 2007 limita esclusivamente a tale componente la possibilità di utilizzo del maggiore gettito (oggi Visco annuncia due nuovi miliardi di maggiori entrate, ma questi vanno incorporati nel DPEF se sono reali e non sono enunciazioni). In ordine alle modalità applicative della nuova disciplina in materia di studi di settore rimane un'incertezza di fondo, un'ambiguità che va superata; appare necessario un chiarimento rispetto agli impegni assunti, con miglioramenti determinati dalla nostra azione relativamente all'onere della prova, alla natura sperimentale degli indici di normalità e agli automatismi. Avete realizzato una politica fiscale vessatoria dovuta alla impostazione assunta dagli studi di settore, passati da strumento di mera selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli a veri e propri metodi di determinazione presuntiva del reddito di tipo statalistico, peraltro senza tenere conto delle scritture contabili, in dispregio del principio costituzionale della capacità contributiva. Va chiarito se tutto ciò sia poi suscettibile di influenzare il livello di gettito acquisibile rispetto a quello preventivato dal Governo. In tema di politica fiscale, sono richiesti interventi incisivi, volti a ridurre il carico fiscale dei lavoratori per i guadagni di produttività e per i premi aziendali.

elevando il reddito effettivamente disponibile delle categorie produttive. Per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, sono necessarie misure volte ad alleviare il carico tributario che grava su questi comparti, come è avvenuto in Germania e in Spagna e come è nel programma di Sarkozy. Una seria politica di contrasto all'evasione fiscale è una ricerca degli evasori e non un sovraccarico sui contribuenti già noti e leali con il fisco. Si rispetti lo Statuto del contribuente; si eviti l'introduzione di norme tributarie con effetto retroattivo, rafforzando l'autonomia del garante del contribuente e dotandolo di adeguate risorse umane e finanziarie. Si proceda per una più forte semplificazione fiscale, riducendo gli adempimenti, evitando circolari chilometriche

Occorre operare una radicale correzione degli indirizzi di politica economica, finalizzandola al rinnovamento del Paese, nel senso di un deciso rafforzamento della sua posizione competitiva e della liberalizzazione di settori e comparti sinora caratterizzati da protezioni e limiti all'accesso di nuovi operatori. È urgente adottare dispositivi di riordino della spesa pubblica in grado di operare il contenimento della componente corrente, mediante una efficace e costante azione di riduzione di quella improduttiva e degli sprechi,

concreto ed efficace, attraverso l'introduzione del principio del contrasto di interesse tra i vari soggetti di imposta, che non è «una balla colossale» come ha affermato il vice ministro Visco.

per le contraddizioni della sua maggioranza, è incapace di operare per il bene del Paese che ha bisogno soprattutto di ridurre la spesa pubblica riqualificandola, La coalizione è paralizzata sulle scelte di investimento per le infrastrutture essenziali (lo abbiamo visto nella relazione del senatore Ripamonti rispetto alle infrastrutture nel Mezzogiorno e sulle direttrici transeuropee)

Signor Presidente farò un breve commento, nei dieci minuti che mi sono consentiti, soprattutto sulla parte fiscale del Documento di programmazione economico-finanziaria, perché è un aspetto che se è importante per quanto riguarda ovviamente le decisioni generali di politica economica, è altrettanto vero che in questo documento gode di un particolare trattamento di scarsa chiarezza e ancora più scarsa determinazione negli obiettivi della maggioranza di Governo. Essendo quella fiscale una questione molto importante che, negli ultimi mesi, nel primo anno di di Governo della maggioranza di centro-sinistra, ha creato gravi problemi e anche altrettanto forti rimostranze da parte di alcune importanti categorie sociali in particolar modo, penso che

di spesa»; «fisco, Visco: studiamo intervento di dimensioni analoghe a quello tedesco»; «Visco: in prossima finanziaria iniziare a ridurre le tasse». Belle cose: ma perché non sono scritte così, in maniera chiara ed esplicita,

voi aumentate la spesa e il decreto sul tesoretto lo dice in maniera assolutamente inequivocabile, al di là di ogni dubbio. A fronte di questo incremento di spesa, provvederete anche, incrementare le entrate e la pressione fiscale. Anche questo, nonostante le dichiarazioni di principio del vice ministro ministro Visco e del relatore,

che si fa, che si dice? Come si fa a dire che si ridurrà la pressione fiscale quando la si è incrementata, quando si sono create spese e aspettative di spesa tali da rendere assolutamente necessario l'incremento della pressione fiscale in futuro?

l'accordo con le forze sindacali sarà quello che andrà bene, e là, in quella sede, si deciderà cosa fare, vale a dire quello che poi è stato fatto in queste ultime ore. Che documento di previsione è

con la finanziaria scorsa e con un Documento di programmazione economico‑finanziaria che va nel senso diametralmente opposto a quello di

speso dei soldi aumentando il rapporto *deficit*-PIL. Per carità, si può arrivare anche al 3 per cento, ma non venite a dire che riducete la spesa pubblica e la pressione fiscale, perché ammettete implicitamente che la vostra strategia

Un anno fa, abbiamo votato un DPEF molto importante; era il primo della legislatura, in qualche modo era un po' il programma della legislatura e, come certamente i colleghi ricordano, poneva

l'attuale ripresa dell'economia, ma non c'è dubbio che se guardiamo agli anni della precedente legislatura, li vediamo caratterizzati da quei due anni di crescita zero: questo è incancellabile. Il terzo obiettivo del Documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso era l'introduzione di elementi di equità in una società caratterizzata da nuove diseguaglianze e da aree di grave disagio sociale sempre più diffuse. Se avete notato, da due anni a questa parte l'ISTAT dedica una parte del rapporto annuale sulla situazione economica del Paese al tema della povertà. Un tema in qualche modo inusuale rispetto a ciò a cui eravamo abituati. Significa che oggi ci sono gravi problemi in pieghe importanti della società italiana e naturalmente queste ci interrogano dal punto di vista della responsabilità politica e sociale, ma anche dal punta di vista della responsabilità economica, per gli effetti che si producono. Questi erano gli obiettivi che ci eravamo dati l'anno scorso. Che cosa è successo di quegli obiettivi? Ad un anno di distanza, credo che possiamo guardare con una moderata soddisfazione alle cose fatte. Intanto, abbiamo sviluppato una iniziativa legislativa molto importante. La voglio richiamare qui dire, sono elementi significativi: non soltanto la legge finanziaria, ma organici provvedimenti di tutela dei consumatori e di introduzione di misure di liberalizzazione in vari settori. Importanti disegni di legge di riforma: ricordo quella dei servizi pubblici locali, il riordinamento delle Autorità, Autorità, il disegno di legge di modernizzazione della pubblica amministrazione; potrei ricordarne altri, per esempio tutti i disegni di legge delega in materia di completamento della riforma del sistema elettrico e di altri importanti sistemi nazionali dei servizi. quindi svolto un'azione anche dal punto di vista legislativo molto significativa. Abbiamo svolto un'azione molto coerente nei campi dell'azione amministrativa. Ricordo la contrattazione per il pubblico impiego, che lega alla trattativa economica la riforma strutturale; ricordo le decisioni di questi giorni, che naturalmente non ho il tempo per discutere, ma gli accordi sulle pensioni e sulla riforma del *welfare* sono elementi importanti di completamento di una strategia che abbiamo delineato un anno fa.

Il lavoro fatto ha avuto dei risultati, si è tradotto nei risultati, sia sul versante della situazione dei conti pubblici, sia sul versante della della situazione della nostra economia, della crescita e dello sviluppo dell'economia. Ricordo due giudizi (li ricordo, naturalmente, come giudizi sommari): il Governatore della Banca d'Italia, nelle sue considerazioni finali, sostiene che l'Italia ha iniziato finalmente a rimettere in ordine la finanza pubblica e ha ripreso a crescere; il presidente dell'ISTAT, presentando il rapporto di quest'anno sulla situazione del Paese, si colloca sulla stessa linea e dice che la ripresa italiana, per quanto moderata, segna il ritorno all'espansione, dopo un quadriennio di stagnazione. Potremmo, naturalmente, dettagliare questi risultati e analizzarli anche nelle loro componenti. A me, per il momento, interessa sottolineare che sono risultati raggiunti. Certo, non è che ci nascondiamo dietro i problemi che continuano a rimanere, dietro alle questioni ancora aperte. Abbiamo la consapevolezza che i risultati che abbiamo raggiunto non ci devono far dimenticare che ci sono tanti problemi strutturali che devono ancora essere affrontati. Li potremmo citare. Abbiamo ripreso lo sviluppo: 2 per cento circa quest'anno, 1,8 e 1,9 previsti per i prossimi anni, ma sappiamo che permane il divario nello sviluppo con gli altri Paesi europei. effetti, abbiamo ripreso una capacità competitiva sui mercati internazionali, ma sappiamo che la nostra quota di partecipazione al commercio mondiale continua a diminuire; quindi, su questi problemi dobbiamo ancora fare un sforzo significativo. vero che la produttività della nostra impresa ha ricominciato a crescere, ma sappiamo che l'anno scorso la produttività delle imprese italiane è cresciuta di un punto, mentre quella delle imprese tedesche è cresciuta di cinque punti, se non ricordo male. Sappiamo, dunque, che ci sono molte questioni strutturali. Le questioni strutturali riguardano anche la situazione dei conti e la finanza pubblica. Abbiamo fatto un'operazione di risanamento sul lato delle entrate. Non è che ci nascondiamo dietro ai dati: sappiamo che ci sono luci ed ombre. Allora, il problema di questo Documento di programmazione economico-finanziaria è riuscire a consolidare e rendere permanenti i risultati raggiunti. Lo dice molto bene il Ministro dell'economia nella lettera di trasmissione del Documento, che rappresenta in qualche misura una buona sintesi degli obiettivi dello stesso, quando afferma che il vero problema che abbiamo di fronte è appunto consolidare e rendere definitivi e permanenti i risultati, in particolare assicurare e garantire una crescita significativa e duratura dell'economia:

ad una situazione in cui tutti gli anni non dobbiamo cercare miliardi di euro per avviare e continuare in un processo di di rientro nei parametri che ci sono stati indicati a livello europeo, ma soprattutto per risolvere il problema del *deficit* dei nostri conti, che costituisce una palla al piede per l'economia. ripeto - lo vogliamo dire in modo chiaro e molto forte: per il 2008, per raggiungere i risultati che ci siamo impegnati a rispettare, nel percorso verso il pareggio del bilancio del 2011, con la

cominceremo domani, non voglio anticipare una discussione che faremo nelle sedi proprie. Personalmente, la considero una buona decisione. Nel suo nucleo fondamentale costituisce un incentivo alla crescita della domanda interna grazie a tutti fa chiarezza sugli impegni sottoscritti, le prassi consolidate, le nuove iniziative come obiettivi da realizzare per i quali viene fatta la scelta di finanziarli con l'aumento della spesa e non con nuove entrate: una coraggiosa azione sul fronte della spesa primaria, che è il vero nucleo centrale rilevante di questo Documento, attraverso strumenti di cui avremo modo di parlare. I colleghi hanno insistito sul tema della riduzione della pressione fiscale: guardate che per noi e per voi il problema non si risolve declamandolo come uno *slogan*,

Documento, che consentirà di affrontare seriamente nei prossimi anni tutti quei problemi che sono stati già richiamati: le infrastrutture, la formazione, la necessità di costruire nuove risorse per un Paese

la comunità degli economisti ha accolto il DPEF con un misto di scetticismo e dure stroncature. «È un documento profondamente sbagliato», ha detto Alberto Alesina. «Illusoria la promessa di una manovra indolore», ha continuato Luigi Spaventa. «Un atto privo di ogni utilità la cui unica funzione è quella di offrire gli argomenti per i primi dibattiti da spiaggia», ha rincarato la dose Nicola Rossi, e potremmo continuare. problema è serio perché queste valutazioni critiche si accompagnano ai giudizi negativi delle più autorevoli istituzioni italiane e straniere: dalla Banca d'Italia alla Banca centrale europea, dal Fondo monetario internazionale all'OCSE.

Ed è su questo che ci si dovrebbe interrogare. Sia nel DPEF, ma soprattutto nella politica finanziaria del Governo, vi sono molti punti oscuri, alcuni evidenti, altri più nascosti. La somma di queste incongruenze alimenta il clima di sospetto e di sfiducia. Iniziamo dai difetti più evidenti. In marzo, con la relazione unificata dell'economia e della finanza pubblica, era stato previsto, per il 2007, un *deficit* del 2,3 per cento. La previsione, comunicata alla Commissione europea, era stata apprezzata. L'Italia appariva quindi come un grande Paese virtuoso che, sfruttando il lascito positivo del precedente Governo, continuava nella strada del risanamento.

Da qui le critiche della Commissione. La previsione di un *deficit* per il 2007 pari al 2,5 per cento è in parte frutto di un artificio. Esso sconta spese di competenza dell'anno in corso, rinviate al 2008. Si tratta, in particolare, di 1,43 miliardi di euro pari allo 0,1 del PIL - corrispondenti ai contratti del pubblico impiego, statali esclusi, ed ai maggiori oneri relativi al personale della scuola. Se queste poste fossero correttamente contabilizzate, il *deficit* effettivo risulterebbe pari al 2,6 per cento: 0,3 punti di PIL in più rispetto a quanto comunicato a Bruxelles ed al lascito del Governo Berlusconi. Non voglio riaprire la questione di chi sia stato il merito del risanamento. Mi limito a ricordare che, nel DPEF del 2001, l'allora ministro del tesoro Vincenzo Visco indicò nello 0,8 per cento del PIL il *deficit* di quell'anno. Alcuni non ci credettero ed avanzarono l'ipotesi di un *deficit* sommerso molto più consistente. L'ISTAT, qualche anno dopo, ne certificò la dimensione indicando un valore pari al 3,1 per cento e quindi fuori dai parametri di Maastricht. Forse memore di quell'esperienza, l'attuale Ministro dell'economia e delle finanze ha cercato di giocare d'anticipo, indicando nello scorso DPEF un *deficit* per il 2006 pari al 4 per cento, che nel programma di stabilità del dicembre 2006 veniva portato al 4,8 A questo risultato si perveniva con una serie di manipolazioni che, per fortuna, i mercati finanziari hanno valutato con un pizzico di buon senso. Se così non fosse stato, il *rating* nei confronti del nostro Paese sarebbe precipitato, con esiti disastrosi. Il *deficit* di base fu ricalcolato per tener conto di quelle maggiori entrate da cui sarebbe nato il "tesoretto", riducendo nello spazio di pochi mesi, da luglio a dicembre, il *deficit* dal 4 al 2,7 Naturalmente queste oscillazioni previsionali non sono senza conseguenza per la credibilità del Paese e ciò si sta ripetendo. Lo confermano le indicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze quando elenca le spese già previste per la prossima legge finanziaria e, almeno per il momento, senza indicazione di copertura, spese che saranno ancora maggiori, considerando l'accordo raggiunto sulle pensioni.

lavoreranno meno ma percepiranno una pensione destinata a decrescere fortemente in termini reali. Le pensioni minori saranno pari al 70 per cento della retribuzione media degli ultimi cinque anni o dieci anni, a seconda che si applichi il metodo retributivo o contributivo.

Le considerazioni appena esposte spiegano il voto contrario del Partito repubblicano. Di questo Governo non apprezziamo la linea di politica economica ed il continuo cedimento alle pressioni della sinistra massimalista.

Abbiamo il timore, però, che su questa linea egli non potrà e non saprà resistere, anche se saremmo lieti di essere smentiti.

e colpevolmente trascurata sia nella relazione del Governo sia nell'illustrazione del relatore. La disparità territoriale mancanza della competitività dei territori nella nostra lunga Italia rappresentano un tema che non viene neanche sfiorato. Il relatore ha fatto delle sottolineature su esigenze

poi come considerare, se non almeno imbarazzante, l'analisi liquidatoria sulle cause del sottosviluppo nel Mezzogiorno. A pagina 105 si dà come unica causa del sottosviluppo - leggo testualmente - «la carenza nella fornitura di beni primari, quali legalità e sicurezza».

la voce disperata di 270.000 giovani che lasciano il Mezzogiorno per raggiungere altre zone dell'Italia. Colleghi della maggioranza, la vostra politica non solo è dannosa per questi territori, ma viene percepita come tale, per cui le nuove generazioni non possono non possono neanche coltivare quella inconsistente ma fondamentale componente dell'emanciparsi che è rappresentata dalla speranza per il futuro. Voi avete ammazzato la speranza dei giovani del Mezzogiorno! Nel Documento di non si intravedono neanche le minime linee guida ed indicazioni per poter superare questo stato di fatalità. Ci avete tolto il ponte, ci avete tolto tutto quello che potevate. Forse volete che la Sicilia ed il Mezzogiorno siano terre di consumatori, dove l'assistenzialismo possa sempre continuare a mantenere una tranquillità sociale, ma non è più questo il tempo non è più questo il tempo e ciò non è più consentibile; noi saremo vigili ed attenti. Mi rivolgo soprattutto alla parte della cosiddetta sinistra radicale della maggioranza, che ha fatto dell'equità sociale una delle bandiere condivisibili nelle linee di principio, per evidenziare che nell'odiatissima America la mobilità tra le classi sociali,

invece, la mobilità sociale è di appena il sei per cento. La mancanza di mobilità sociale viene attribuita a due fattori fondamentali: la mancanza di liberalizzazioni e la mancanza di un efficace sistema di formazione e di cultura. Bene, questo DPEF uccide, nel senso che non propone soluzioni allo stesso tempo sia per l'uno che per l'altro aspetto, perché non ci sono vere liberalizzazioni e perché ancora una volta non considerate strategica la formazione; ancora una volta tagliate fondi per l'università e la ricerca e ancora una volta non dite una parola su cosa dovrà fare da grande il nostro Paese. Sembra un vivere quotidiano alla rincorsa di compromessi sempre a più basso livello. Per garantirvi la governabilità, si dovrebbe dire; purtroppo, però, è soltanto

la sostanziale condivisione della relazione del senatore Ripamonti, da lui integrata oralmente oggi in Aula, mi consente di dare un taglio esclusivamente politico a questo mio intervento. Il DPEF fotografa l'economia italiana in ripresa sostenuta. I risultati complessivi permettono, tra l'altro, una prima azione redistributiva, quella contenuta nel decreto extragettito, che sarà alla nostra attenzione la prossima settimana. È la conferma di una nostra previsione, che ci aveva indotto a chiedere - a noi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - l'anno scorso, di spalmare su due anni gli interventi atti a sistemare i conti pubblici, senza disattendere con questo le sollecitazioni dell'Unione Europea. Fosse stata accolta quella nostra proposta, forse oggi il clima sociale nel Paese sarebbe migliore. La ripresa, che si inserisce in una fase di crescita globale, poderosa e e destinata a continuare, anche se non vanno sottovalutati i segnali in controtendenza, è stata alimentata in gran parte dalla domanda interna e ha avuto come volano un sistema produttivo che si è ristrutturato: il caso FIAT è emblematico. Il Governo di suo ha messo un rinnovato vigore nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, con buoni risultati; un maggiore rigore nel monitoraggio della spesa pubblica e nella sua erogazione, anche se con alcune forzature tecniche, non sempre comprensibili, non sempre condivise. Ha messo un'attenzione intelligente al rifinanziamento di cantieri e opere pubbliche, anche se non tutti i risultati sono stati pari alle attese. È evidente che il Paese ha un problema serio rispetto alle proprie vie di comunicazione, al trasporto delle merci e delle persone. Ferrovie, trasporto aereo, autostrade del mare, riduzione dell'incidenza dei vettori gommati sono temi decisivi per un Paese che aspira ad una modernizzazione compatibile con i nuovi scenari demografici, ecologici, economici, urbani e sociali che si stanno delineando. Il Governo lo scorso anno ha chiesto altri sacrifici al Paese, pur intraprendendo un timido tentativo di redistribuzione, agendo sulla rimodulazione delle aliquote fiscali. Oggi è ora di cambiare passo. «Se non ora quando?», uno *slogan* che ha utilizzato anche il collega Tecce in Commissione. Noi non concordiamo con chi sostiene che è in periodi di crescita che si deve procedere con più convinzione ad aggiustamenti strutturali, perché così si esclude qualsiasi possibilità di una vera redistribuzione della ricchezza prodotta dal Paese, essendo chiaro che durante le crisi le politiche espansive non sono facilmente praticabili. Da qui la vera sfida che proponiamo al nostro Governo: impegnarsi perché in una fase di forte crescita economica a trarne beneficio siano prima di tutti i lavoratori, i precari, chi si ama e vuole vivere sotto lo stesso tetto, i pensionati, insomma coloro che hanno sempre stretto la cinghia e che continuano a farlo, che hanno - se mi si concede una pennellata veltroniana - rinunciato ai loro sogni. Non ci facciamo facili illusioni. Sui temi del lavoro stiamo registrando la possibilità di una rottura. La difficoltà è vera, è grave, perché rimanda prima di tutto ad una divaricazione delle culture politiche delle forze della coalizione. La faticosa, ma seria ed efficace sintesi del programma dell'Unione è in discussione, può finire a pezzi. Ma nel DPEF è descritto un Paese, sono delineati scenari finanziari, economici e sociali favorevoli ad una ricomposizione in nome dell'equità e della redistribuzione, senza dovere rinunciare ad un'impostazione da *civil servant* nella gestione dei conti pubblici. Vedremo se la nostra attività legislativa futura saprà cogliere questa occasione. Certo, a legislazione vigente non avremmo bisogno di alcun intervento per la correzione dei conti. È una buona notizia. Ma a legislazione vigente, il Paese in cui viviamo non è il miglior Paese possibile: è la verità. Al di là della sua quantificazione, e prestando la massima attenzione agli equilibri finanziari, è evidente che la manovra lorda, cioè l'insieme dei nuovi interventi da realizzare nel 2008, è la leva che abbiamo a disposizione per quel cambiamento di passo necessario

Siamo convinti che già nella risoluzione della maggioranza alcune linee guida, qui sommariamente indicate, possano ritrovarsi e condurre questa coalizione a quel cambiamento di passo a cui ho accennato.

il gravissimo aumento della pressione fiscale attuato dal Governo Prodi in poco più di un anno, che sta avendo ed avrà un pesante effetto di rallentamento dello sviluppo del Paese.

uno spaventoso aumento del 2,2 per cento, frutto di una concezione radicale e insensata del bipolarismo, assolutamente insostenibile per il Paese. Gli italiani ricorderanno. Dedico i pochi minuti a mia disposizione all'esame della politica energetica. Per quanto riguarda le linee generali di tale politica, così importante per un'economia di trasformazione come quella italiana, notiamo le stesse carenze già rilevate nel DPEF 2007-2010: nessuna iniziativa incisiva per diminuire il troppo elevato costo del chilowattora, anzi esclusione di qualunque menzione dell'energia nucleare e nessun accenno al possibile importante ruolo del carbone; solo declamazione di ovvietà sui benefici di una maggiore concorrenza e sulla necessità di impianti rigassificatori e di nuovi gasdotti. Circa il complesso problema dei cambiamenti climatici in atto e delle loro cause, constatiamo la totale mancanza di qualunque autonomia di pensiero. La linea è quella dell'IPCC, che attribuisce il riscaldamento globale in atto all'anidride carbonica antropogenica. Una linea ancora molto discussa in sede scientifica. E anche in qualche modo contraddetta dallo stesso IPCC, quando fornisce per varie attività umane aventi effetto sul clima (come l'agricoltura, la deforestazione e la produzione di aerosol) valori dei *forcing* radiativi confrontabili con quello dell'anidride carbonica. Gravemente inadeguata è la presentazione dei problemi derivanti dall'applicazione del Protocollo di Kyoto. Non vi è il benché minimo accenno al fatto che le regole di applicazione del Protocollo (colpevolmente sottoscritto a suo tempo dal Governo di centro-sinistra) penalizzano ingiustamente il nostro Paese, in cui la produzione termoelettrica, basata in gran parte sulla combustione di gas naturale in moderni impianti a ciclo combinato ad alto rendimento, è la meno inquinante di tutti i Paesi dell'Unione Europea, in termini di tonnellate di anidride carbonica per megawattora prodotto. Nel paragrafo "Clima e ambiente" si accenna all'obiettivo comunitario assunto dal Consiglio europeo di primavera, consistente nella riduzione dei gas serra all'80 per cento di quelle del 1990, entro il 2020. L'obiettivo è per il nostro Paese totalmente irraggiungibile, non essendoci ormai più quasi nessun margine di miglioramento delle emissioni di gas serra nel settore termoelettrico. Diventa quindi decisiva la linea del Governo nel negoziato per l'ormai prossimo *burden sharing agreement* riguardante questo obiettivo. Ma di tale linea non vi è alcuna traccia nel Documento al nostro esame. Per far fronte all'obiettivo, l'unica possibilità prospettata nel DPEF è quella di un «deciso aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili». Non viene detto però come potrà essere realizzato questo aumento. L'energia idroelettrica è ormai in saturazione e per di più la siccità di questi anni ne diminuisce il contributo. Anche per l'energia geotermica non si prevedono importanti aumenti. Le uniche fonti rinnovabili suscettibili di un certo incremento sono l'energia eolica e l'energia da biomasse. Ma per tanti motivi non potremo certamente avere nel nostro Paese lo sviluppo dell'energia eolica che si è avuto (e che si sta avendo ancora) in altri Paesi europei, come la Danimarca, la Spagna e la Germania. Manca inoltre nel DPEF un qualsiasi accenno ad una fonte energetica (da considerarsi parzialmente da biomasse) che nel resto d'Europa dà un contributo non trascurabile alla produzione di energia elettrica: la combustione dei rifiuti solidi urbani. Non si tratta di una banale dimenticanza, ma dell'espressione di una linea di ambientalismo radicale, purtroppo prevalente nel Governo Prodi. Una novità assolutamente negativa, a nostro avviso, è quella della previsione dell'estensione del finanziamento in conto energia all'energia elettrica prodotta da fonte solare termodinamica a concentrazione, per cui si prospetta la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di almeno 500 MW di energia elettrica. Il finanziamento in conto energia è, in sostanza, una forma di tassazione a carico degli utenti degli utenti del sistema elettrico, in cui l'esazione avviene mediante la voce «A3» della bolletta elettrica, già applicata per l'assurdo finanziamento dell'energia elettrica fotovoltaica, con un onere complessivo di 13 miliardi di euro. Tra le fonti rinnovabili un altro miraggio del DPEF è quello dell'agroenergia. Al riguardo Al riguardo sappiamo bene come stanno le cose. Nel caso più favorevole per le produzioni agricole italiane (quella della barbabietola da zucchero) si possono al massimo ricavare per anno e per ettaro 6 metri cubi di etanolo, equivalenti a 3 tonnellate di petrolio. A parte l'insostenibilità l'insostenibilità economica di tale produzione, il contributo di questa fonte energetica al nostro fabbisogno annuo di petrolio non potrebbe che essere estremamente modesto: un milione di ettari, cioè 10 mila chilometri quadrati, coltivati a barbabietola, produrrebbero non più del 3 per cento del nostro consumo annuo di petrolio! In conclusione, il DPEF 2008-2011 risulta sulla politica energetica, essenziale segmento della politica economica, privo di vera capacità propulsiva, incapace di affrontare i gravi problemi strutturali della realtà del nostro Paese, sostanzialmente bloccato dalle drammatiche divergenze ideologiche esistenti all'interno della coalizione di centrosinistra al Governo.

il *fil rouge* che lega tra loro le diverse parti del DPEF 2008-2011 è la volontà di assicurare lo sviluppo economico attraverso interventi sostenibili: dal punto di vista degli equilibri di bilancio, dell'equità sociale e della compatibilità ambientale. Un documento e degli obiettivi credibili, perché viene prestata la dovuta attenzione al reperimento delle risorse. Si esclude un ulteriore aumento della pressione fiscale (la quale, anzi, è destinata a ridursi), i finanziamenti sono ricercati altrove: principalmente nella lotta all'evasione, con positivi riscontri anche sull'equità sociale e sul corretto funzionamento del mercato; nella razionalizzazione della pubblica amministrazione, con ciò che ne deriva anche in termini di miglioramento dei servizi alla comunità, di avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, di competitività per le aziende. Il tutto, poi, si innesta sul nuovo progetto in *itinere* di un'Italia rinnovata nelle sue articolazioni e nei suoi rapporti interni, sulla base dei disegni di legge di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione: il cosiddetto codice delle autonomie e il federalismo fiscale (con l'auspicio che sia un vero federalismo fiscale). La complessità del quadro è di tutta evidenza, ma credo che il percorso sia ben tracciato. La conferma dovrà avvenire, chiaramente, in prima battuta, sin dalla prossima legge finanziaria. Poi si dovranno monitorare i risultati delle iniziative previste, una volta avviate. Due richiami di carattere generale. Primo: la razionalizzazione della spesa. Dev'essere calibrata, mirata, ben fondata su solidi presupposti. Razionalizzare non significa produrre risparmio a discapito del servizio, ma spendere meglio. Occorre ottimizzare il risultato, passando anche attraverso adeguate economie. Nel caso contrario il rischio è quello di erodere il meccanismo pubblico sino ad un livello critico, di non essere pronti ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità della crescita economica, di accrescere le differenze interne. Il secondo richiamo riguarda le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, che devono vedere rispettati e valorizzati, in ogni momento, i loro ambiti di autonomia. Ogni scelta, ogni decisione, dev'essere partecipata: a salvaguardia delle rispettive competenze e quale garanzia essenziale per il successo delle azioni. Sono confortanti le previsioni sulla crescita, sul riequilibrio della finanza pubblica, sulla riduzione della disoccupazione. Ho cercato di leggere il Documento in una logica "pratica", di rapporti tra cittadino, imprese e istituzioni e tra i diversi livelli di Governo, ricercando quei vantaggi competitivi in grado di fornire alimento alla costruzione di un'Italia più solida e partecipata, rispettosa delle differenze, quindi di un'Italia più giusta e in grado di colmare i divari, attraverso approcci diversi per situazioni diverse. Da qui, alcune osservazioni. Giustizia, legalità e sicurezza: la loro efficienza è parametro della civiltà di un Paese; la loro efficacia è garanzia della credibilità delle istituzioni. Investire in questo settore è vitale: per lo sviluppo economico e per lo sviluppo civile. La legalità dev'essere cultura e valore. La sicurezza dev'essere soprattutto prevenzione e azioni in favore della "sicurezza percepita" dai cittadini, della sicurezza "partecipata" da tutti i settori della società e da tutti i livelli di governo. Opportuna una corretta politica volta ad ottimizzare i servizi e a promuovere una cultura realmente orientata al mercato. Le peculiarità dei diversi territori non possono tuttavia essere ignorate, e quelle dei territori di montagna in particolare. Per quanto concerne, per esempio, il servizio postale, dev'essere ovunque mantenuto a livelli adeguati e rispondenti alle esigenze della popolazione. Clima, ambiente, energia: tre altre grandi priorità del nostro tempo. Credo sia essenziale realizzare attività di educazione all'ambiente e al risparmio energetico: per favorire il sorgere di una cultura orientata verso tali obiettivi, più efficace di qualsiasi norma e di qualsiasi coercizione. Nel settore "politiche del lavoro", di rilievo sono gli obiettivi della lotta al sommerso e al lavoro irregolare, alla sicurezza e salute dei lavoratori, ma soprattutto l'aver centrato le criticità che toccano le donne, i giovani e i lavoratori *over* 50. La scuola, l'università, la ricerca. Qualità, programmi adeguati alle necessità del mondo del lavoro, ricerca di sinergie tra le università e le imprese: sono esigenze imprescindibili. Come lo è garantire il diritto allo studio per i nostri giovani, in ogni parte del Paese, attraverso una capillare presenza degli istituti e il loro mantenimento nei territori di difficile accessibilità Condivisibili le linee tracciate in ambito di equità sociale e di semplificazione del sistema tributario. Un appunto sulla cooperazione allo sviluppo. È necessaria una maggiore apertura, bisogna lasciare più spazio alle Regioni e Province autonome, se si vuole fare della vera cooperazione: profonda, in grado di saldare rapporti di fiducia e di amicizia tra persone e popoli diversi. Urge riconoscere il ruolo della cooperazione decentrata, con il solo limite della "non incompatibilità" con la politica estera dell'Italia. Ancora tre argomenti di riflessione: le minoranze, le autonomie differenziate, la montagna. Il DPEF avrebbe forse potuto essere più incisivo: ne è carente. Le diversità "positive", quelle che aggiungono un *plus* alla nostra Repubblica, devono essere rispettate, salvaguardate, valorizzate, siano esse istituzionali, culturali, territoriali. Mi ha colpito la previsione di un Fondo volto a valorizzare e promuovere le realtà socio-economiche delle zone di confine tra le Regioni a Statuto ordinario e quelle a Statuto speciale, al fine di disincentivare il fenomeno dei distacchi dei Comuni. Le autonomie differenziate vengono viste quasi come un elemento di disturbo, semplicemente perché, con la loro autonomia, hanno saputo fare sviluppo. Non ci si può dimenticare i fondamenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome e della loro autonomia finanziaria, che devono continuare ad essere integralmente garantiti. Forse, una scelta più coerente sarebbe l'attribuzione di più autonomia per tutti. la montagna, è necessario procedere rapidamente e in termini globali, come previsto dal disegno di legge n. 1607. La montagna è patrimonio, culturale, ambientale, energetico, da salvaguardare e da valorizzare. Siamo spesso confrontati a norme ed iniziative che in qualche maniera inglobano i tenitori di montagna tra le aree disagiate in generale, senza riconoscerne le peculiarità. Necessario, invece, riconoscerle, queste specificità, perché la montagna è strutturalmente diversa. Ha costi superiori. Il territorio è sensibile e dev'essere mantenuto, deve rimanere antropizzato anche a vantaggio delle pianure. Fornire alla montagna gli strumenti per vivere è investire in qualità e per prevenire le catastrofi naturali e i costi che queste comportano. È riconoscere il dovuto a popolazioni che rischiano di essere espropriate della loro cultura e delle loro risorse, in nome degli imperativi del mercato. Nella sostanza, ciò che più serve è riconoscere alla montagna la sua diversità; è riconoscerle il diritto di sottostare a regole diverse, in grado di sviluppare le sue potenzialità sulla base di linee di governo e di sviluppo condivise dagli stessi montanari. Infine, apprendo con soddisfazione che il programma delle infrastrutture allegato al DPEF contempla le esigenze a più riprese segnalate dalla Regione Valle d'Aosta, sempre in un obiettivo di sviluppo e di apertura correlato alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza della circolazione. Si tratta di interventi che permetteranno una maggiore coesione territoriale e una migliore integrazione commerciale dell'Italia con il resto dell'Europa. Sono tutti interventi attesi da tempo, urgenti, la cui realizzazione dev'essere garantita dalla necessaria copertura finanziaria che, si confida, sarà adeguatamente assicurata dal Governo. Soddisfazione, anche, per l'aver rispettato le pronunce del consiglio regionale della Valle d'Aosta, contrarie ad un eventuale raddoppio del Traforo del Monte Bianco. La garanzia del Governo su questi punti - ruolo delle Regioni e degli enti locali, autonomie differenziate, minoranze, montagna, infrastrutture - è condizione per un parere favorevole sul Documento.

il Documento di programmazione economico-finanziaria conferma nei dati la validità delle scelte che sono state fatte in quest'anno di Governo. Quello che ha funzionato è stato il tenere strettamente legati gli obiettivi di risanamento, di crescita e di equità. Quindi, quando il senatore Vegas parla di lubrificazione della spesa sociale per sostenere il consenso, nel migliore dei casi non ha presente che il nostro Paese, rispetto al resto dell'Europa, ha una situazione di debolezza del sistema che è determinata, oltre che da una bassa capacità di innovazione, dall'inefficienza della pubblica amministrazione, dalla penuria di infrastrutture, da un alto livello di povertà che ancora tormenta le famiglie, da una partecipazione molto più bassa che nel resto d'Europa delle donne al mondo del lavoro e, infine, da un basso grado di istruzione della nostra forza lavoro. Di conseguenza, il raggiungimento di una crescita più alta dipende anche da un maggiore coesione nonché da una maggiore equità sociale. Quindi, nessuna lubrificazione ma un'azione coerente per dare solidità e trasformare la crescita da un fatto congiunturale a un fatto strutturale. Nel Documento si sottolinea che i tempi sono maturi per completare lo Stato sociale. Penso che sia particolarmente valido, come sottolineato, per l'aspetto pensioni e sanità, ma non adeguato ai mutamenti che si sono determinati con la globalizzazione, in seguito al saldo demografico negativo e anche per quello che riguarda l'aumento delle persone anziane e dell'immigrazione. Il punto, quindi, è come passare da un *welfare*, che gli studiosi definiscono mediterraneo, a un *welfare* di tipo europeo, che sia basato sull'opportunità e sui diritti, sulla prevenzione e non sull'emergenza. Mi sembra che l'accordo sindacato‑Governo di questi giorni sia un segnale nella direzione di costruire un *welfare* che abbia alla base una maggiore equità intergenerazionale. Però, di fronte alla perdita di forze attive del mercato del lavoro come conseguenza del calo demografico, il tema di una maggiore occupazione femminile non è solo una questione di pari opportunità, ma anche il tema dell'apporto concreto che noi pensiamo di poter dare al sviluppo della ricchezza del Paese. Per questo colgo in modo particolarmente favorevole l'impegno di una forte diffusione dei servizi, in particolare quelli alla prima infanzia. È infatti nei primi anni di vita del bambino che la maggiore parte delle lavoratrici abbandonano il loro posto di lavoro. Colgo l'occasione per chiedere, tra l'altro, che questa Assemblea metta all'ordine del giorno l'approvazione di un testo per la costruzione della rete dei nidi e dei servizi, perché, oltre all'impegno triennale per la costruzione delle strutture, come è stato previsto nell'ultima finanziaria, occorre una legge per sostenere i costi di gestione, che oggi ricadono interamente sui Comuni, e per sostenere le rette che vengono pagate interamente dalle famiglie. Le risorse potrebbero essere trovate in un'adeguata riorganizzazione della spesa per l'istruzione primaria. Infine, quello della qualificazione della spesa è proprio uno degli obiettivi che si pone il Documento di programmazione economico-finanziaria, quindi è importante che questo venga fatto anche nella direzione di trovare nuove risorse per nuovi investimenti nel campo dei servizi. È importante anche che l'attenzione sia rivolta agli anziani non autosufficienti e trovo che sia importante che quanto prima vengano definiti, così come indicato nel Documento, i livelli essenziali di assistenza in questo settore e poi costruire un patto con le Regioni per favorire una loro compartecipazione alla spesa. Mi consenta, Presidente, di riferirmi brevemente anche a quello che riguarda la parte di programmazione in campo sanitario. Ritengo che l'impegno e l'ammodernamento del sistema sanitario sia oggi uno degli elementi necessari per, innanzitutto, valorizzare le risorse umane, il superamento del precariato, l'innovazione tecnologica e, infine, anche la possibilità di riorganizzare tutto il sistema di cura, partendo dalle cure primarie, proprio a sostegno dell'attenzione verso le malattie croniche che oggi tormentano una grossa parte della nostra popolazione anziana. Consentire la continuità di cura dev'essere uno dei nostri obiettivi e a questo scopo mi pare molto importante anche sostenere l'integrazione socio-sanitaria, soprattutto nel momento in cui chiediamo una collaborazione ai Comuni per integrare l'assistenza sanitaria sul territorio. Infine, importante è questo sforzo d'adeguamento dell'edilizia sanitaria, sia questa ospedaliera o di

a quella sulla stessa utilità di mantenere questo strumento, il DPEF appunto. Ciò è dipeso dalla circostanza che talvolta ci siamo trovati a discutere di documenti che non avevano nessuna delle caratteristiche degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, spesso presentati in ritardo, poco chiari, incompleti, confusi, omissivi e reticenti, spesso in evidente contraddizione con i processi economici nazionali e internazionali e con il Paese reale. Quest'anno deve essere riconosciuto innanzitutto al Governo di aver presentato al Parlamento nei tempi previsti un Documento che ha il merito della completezza, della chiarezza, un contributo alla trasparenza al servizio di un'operazione "verità", di cui il Paese aveva bisogno. Ci troviamo altresì in presenza di un nuovo sistema di classificazione del bilancio, che rende il bilancio più trasparente e più comprensibile ai cittadini e al Parlamento. Il Documento di programmazione economico-finanziaria non è pertanto lo strumento da utilizzare per la propaganda - voglio tranquillizzare il collega Vegas -, come spesso è stato, questo sì, nel passato, ma per fotografare il Paese reale e indicare linee di politica economica e sociale da tradurre in provvedimenti legislativi, a partire dalla legge finanziaria, coerenti con il programma elettorale e con gli interessi e i bisogni veri e concreti dei cittadini e del Paese. Il Documento di programmazione economico-finanziaria al nostro esame parte quindi dalla constatazione che gli sforzi per il risanamento sono già stati in larga misura fatti. Il DPEF quindi opta per un percorso veramente rigoroso ma più graduale, che coniuga l'esigenza di utilizzare una gran parte delle risorse aggiuntive emerse nel 2007 a riduzione del disavanzo, al fine di evitare una nuova manovra correttiva nel 2008, con quella di fronteggiare emergenze produttive e istanze sociali di grande rilievo. Quest'anno, come richiamato dallo stesso Ministro dell'economia, prevarranno dunque nella definizione dei provvedimenti da assumere le misure per la crescita e quelle per l'equità sociale. La correzione del *deficit* tendenziale a legislazione vigente per il 2008 non ci sarà, come non si ravvisa la necessità (per la prima volta dopo tanti anni) di una manovra correttiva in corso d'anno per il 2007. Queste priorità sono state rese praticabili da due fattori: un gettito tributario strutturale maggiore del previsto; una rimodulazione della dinamica di riduzione del rapporto *deficit*/PIL possibile grazie ai risultati conseguiti nel corso del 2007. In Italia, dopo un quinquennio di crescita modesta, nel 2006 è iniziata una ripresa economica: è cresciuta l'occupazione; è cresciuta, dopo una preoccupante fase di stagnazione, la produttività del lavoro; segnali positivi provengono dall'andamento delle esportazioni; la produttività totale dei fattori non decresce più, anche se cresce poco in conseguenza della rigidità dei nostri mercati. Per far sì che questa ripresa congiunturale diventi duratura e sostenibile è necessario che il Governo continui il processo delle riforme con determinazione (molte delle quali sono all'esame del Parlamento: la «Bersani 2», la legge sui servizi pubblici locali, l'*Authority*, l'energia, il gas), coniugando crescita economica con equità sociale, risanamento finanziario e sostenibilità ambientale. Questa impostazione del DPEF è stata resa possibile grazie ai risultati conseguiti nel primo anno del Governo Prodi. Si è rifiutata la logica dei due tempi. L'azione di Governo non solo è riuscita nel risanamento dei conti pubblici, ma ha avviato provvedimenti per la crescita e la competitività del nostro sistema Paese e l'equità sociale. Voglio ricordare l'avvio della politica delle liberalizzazioni a favore dei consumatori e degli utenti; i risultati della lotta all'evasione fiscale dopo anni di permissivismo; i provvedimenti sugli assegni familiari, sulle pensioni basse e per agevolare, in maniera ancora certamente insufficiente, i giovani sul terreno previdenziale. Si è iniziato a stabilizzare i lavoratori precari, ad iniziare da quelli delle pubbliche amministrazioni, decine di migliaia, in particolare nella scuola. Infine, voglio ricordare le misure previste nel decreto-legge n. 81 che finalizzano l'extragettito di 6,5 miliardi di euro per il 2007 a misure per la crescita e il sociale. Ovviamente, si può e si deve fare meglio e di più, già a partire dalla prossima finanziaria, ma mi è sembrato giusto ricordare alcuni dei risultati conseguiti. Molti critici sottolineano (lo ha fatto oggi il senatore Vegas) il fatto che le indicazioni del DPEF non rispetterebbero gli impegni del Patto di stabilità: ciò non è assolutamente vero, anzi, è vero il contrario. Il DPEF 2008 rispetta a pieno non solo i parametri dal Trattato di Maastricht, ma anche la raccomandazione dell'ECOFIN del luglio 2005, l'unico documento impegnativo per il Governo italiano. Non solo gli obiettivi programmatici del DPEF rispettano a pieno gli impegni definiti nella raccomandazione ECOFIN per gli anni 2007, 2008 e 2009, ma migliorano in misura notevole l'impegno di ridurre il *deficit* per il biennio 2010-2011. Certo, nessuno può disconoscere il problema di uno *stock* del debito così rilevante per i nostri conti pubblici, tanto più in presenza di una tendenza dei tassi alla crescita con relativo aggravio del servizio del debito. Non è un caso che il DPEF indichi la spesa per interessi tendenzialmente stabile dal 2008 al 2011, malgrado la minore incidenza del debito. Ma non è solo il volume assoluto del debito (ci teniamo molto ad affermarlo) il dato sul quale soffermarci. Dobbiamo anche considerare il suo rapporto con il prodotto interno lordo. L'obiettivo dev'essere, infatti, quello di diluire il debito con la crescita. Ci vuole equilibrio tra questi due parametri: la diminuzione assoluta dello *stock* del debito e la crescita del PIL. Una visione invece unilaterale non può che essere dannosa per il Paese. Schematizzando, il nostro Paese ha quindi davanti a sé due possibilità: la riproposizione del vecchio modello di sviluppo; oppure la scelta della qualità: dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione, della ricerca, della riqualificazione del nostro terziario e del nostro sistema di *welfare* (visto anche come occasione per creare nuovi posti di lavoro), la scelta dello sviluppo della domanda interna pubblica e privata, della buona occupazione. Noi evidentemente scegliamo la strada della qualità e della sostenibilità. Su questo, il DPEF e la risoluzione che sarà presentata sono abbastanza chiari. Non esiste dunque una sola possibilità: lo sviluppo sostenibile per le persone e per l'ambiente è la strada da imboccare, partendo dalla valorizzazione del lavoro e, quindi, in primo luogo, dal rifiuto della logica che presiede alla scelta di rapporti di lavoro privati di dignità e diritti e per questo precari. Vorrei parlare infatti della qualità dell'occupazione, in particolare di quella dei giovani. Si è tanto parlato di dare meno ai padri e più ai figli. In realtà, molti di coloro che sostengono questa tesi vogliono dare meno ai padri e niente ai figli. Se effettivamente si volessero migliorare le pensioni future dei giovani, si dovrebbe agire oggi, da subito, eliminando la precarizzazione del lavoro a cui sono costretti quasi tutti i giovani. Ci sarebbero più contributi, più certezze per la loro vita, pensioni future più alte; al riguardo non si è fatto ancora quanto è necessario. Per queste ragioni critichiamo il Protocollo presentato dal Governo sulla competitività e il mercato lavoro. Una critica di fondo che facciamo alla sua impostazione è che si ispira ad una logica secondo cui una maggior competitività si ottiene con il perseguimento dell'abbattimento del costo del lavoro. Questa è l'idea del lavoro che noi consideriamo sbagliata. I provvedimenti sulla competitività, nel momento in cui, per esempio, defiscalizzano lo straordinario, e cioè fanno costare un'ora di straordinario esattamente come un'ora di lavoro normale, tengono più conto delle esigenze di Confindustria, anche dal punto di vista culturale, piuttosto che di contrastare la precarietà e di proporre un'idea di lavoro di qualità. È evidente che non è questo il modo con cui si aumenta l'occupazione dei ragazzi e delle ragazze. A proposito del lavoro precario, vogliamo fare esattamente quello che è scritto nel programma dell'Unione, per questo ci batteremo e ci siamo battuti fin dalla

in meno; l'occupazione nel Paese cresce dell'1 per cento, mentre nel Mezzogiorno solo dello 0,7; il PIL per abitante nel Mezzogiorno è quasi la metà di quello del resto del Paese;

trasferimenti stabili, la nuova immigrazione tra il Sud e il Nord del Paese; gli irregolari al Sud crescono di 43.000 unità e in tutto sono 1,4 milioni. L'ultimo rapporto dello Svimez ci ricorda, quindi, che le prospettive per il reale avvio di un processo di accelerazione di sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno sono legate al superamento di alcuni vincoli strutturali che hanno impedito all'economia del Sud di reagire positivamente ai colpi provenienti dal nuovo contesto competitivo internazionale. Ovviamente non possiamo sviluppare in questa sede un'analisi approfondita sulle esigenze del Sud, ma abbiamo insistito perché nella risoluzione fossero contenuti alcuni elementi che riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno, a partire dalla rimodulazione delle spese previste nell'Allegato infrastrutture per in quinquennio 2008-2012, in maniera tale da garantire già dal prossimo triennio 2008-2010 una massa reale di investimenti per le opere pubbliche del Sud superiore al 30 per cento di tutti gli investimenti previsti per il Paese. Infatti, l'Allegato infrastrutture rinvia al 2012

Infine, dobbiamo dare il buon esempio a partire dai costi impropri della politica. Si può e si deve fare di più rispetto a ciò che dispone il disegno di legge che stanno predisponendo i ministri Santagata e Lanzillotta che prevederebbe a regime - così come riferiscono gli organi di stampa - risparmi per 1,3 miliardi. Noi pensiamo che si possa arrivare, in una prima fase, almeno a due miliardi di euro di risparmi a regime, chiarendo che dobbiamo tagliare gli sprechi e i privilegi, non i finanziamenti e i costi per garantire una corretta vita democratica del nostro Paese. E chiediamo che i risparmi previsti siano computati fin dal 2008 nella manovra di bilancio destinata a spese di carattere sociale. Sono queste alcune delle ragioni - quante è possibile illustrarne nel tempo che ci è concesso - che ci consentono di apprezzare il Documento proposto dal Governo, di condividere la relazione del relatore di maggioranza e quindi di dare il nostro positivo contribuito ad una risoluzione

Il DPEF conferma sostanzialmente gli impegni assunti nella finanziaria 2007 e apre alla possibilità di un aumento della spesa in conto capitale per il Mezzogiorno e per le infrastrutture. Ma il punto fermo su cui dovremmo interrogarci e su cui chiedo, anche magari nella risposta del Governo,

l'attenzione che la classe dirigente dà al Mezzogiorno è ben più ampia. Ora, il punto è il seguente: queste imprese pubbliche, che agiscono quasi da privati secondo la logica di mercato, possono essere assolutamente estranee e risultare sottratte all'indirizzo politico? Bene si fa, nella risoluzione di maggioranza, a dire che il Governo deve spendere non meno del 30

perché purtroppo ci sono opere già avviate che si devono concludere, ma nel *trend* complessivo noi dobbiamo andare ampiamente oltre al 30 per alla fine, poi, le infrastrutture le fanno l'ANAS e le Ferrovie, e se analizzate il piano strategico delle Ferrovie nel Sud

n. 488 nel credito d'imposta per l'occupazione. Tale legge, negli ultimi anni, ha incontrato grandi difficoltà burocratiche: ci sono stati circa 6.000 accertamenti della Guardia di finanza le imprese hanno trovato grandi difficoltà. Occorre sostituire quella legge con il credito di imposta sull'occupazione. Questo darebbe maggiore trasparenza

rimasto). Per la prima volta, con la finanziaria del 2007, abbiamo armonizzato il fondo per le aree sottoutilizzate con i fondi europei, creando condizioni di certezza finanziaria per il periodo che va fino al 2015, perché si tratta di circa 100 miliardi di euro per il Mezzogiorno

è un progetto organico sul Mezzogiorno. Il quadro strategico nazionale non è sufficiente, perché individua solo una serie di parametri, una serie di percentuali.

non dico completamente ma almeno in parte, il Nord e a diminuire il divario che separa il Nord dal Sud, saremo condannati ad un dualismo strutturale incancellabile per il Paese.

Nella manovra economica e finanziaria dello scorso anno c'era quasi una cesura tra le misure di risanamento e di razionalizzazione e gli obiettivi di crescita della scuola, dell'università e della ricerca, che pure in quella manovra erano contenuti. Il DPEF al nostro esame, da questo punto di vista, è un passo avanti e può essere preludio ad una finanziaria che dia risposte positive a tali problematiche. affermata la necessità di un legame stretto tra misure di razionalizzazione e misure volte ad aumentare i livelli più generali di istruzione e di formazione delle persone, incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione. C'è l'impegno a reinvestire nella scuola, nell'università e nella ricerca gli eventuali risparmi in una logica di incremento del peso che le politiche del sapere devono avere nelle scelte più complessive di politica economica e sociale del Paese. Del resto, lo stesso rapporto OCSE sull'Italia

che con più decisione sono entrati nell'economia e nella società della conoscenza. In particolare, l'OCSE afferma che la scarsa rotazione di capitale umano e la scarsa capacità del nostro sistema economico e produttivo di utilizzare il capitale umano, i talenti e i meriti, è una delle ragioni di fondo per cui l'Italia a livello di produttività e competitività cresce meno degli altri Paesi europei. Guardate, però, che non c'è solo una ragione economica, c'è anche una ragione sociale perché, se c'è un limite nell'apprezzabile, giusto, corretto accordo sulle pensioni, se c'è un limite nello stesso Documento sul *welfare* che il Governo ha presentato alle parti sociali, è ancora la scarsa attenzione che le politiche della formazione hanno nel ridisegnare un nuovo *welfare* delle promozioni dell'opportunità rispetto ad un *welfare* di puro risarcimento. Lo stesso relatore affermava che la sostenibilità del sistema pensionistico in un Paese in cui è drammaticamente basso il tasso di occupazione delle persone sopra i si basa su politiche di invecchiamento attivo, perché finché in questo Paese le persone sopra i 55 anni che lavorano sono il 39 per cento della popolazione, contro il 69,2 della Finlandia, della Svezia e di altri Paesi, non c'è nessun sistema pensionistico che alla lunga regga.

per riprendere un discorso che finalmente dia valore alla cura delle persone che lavorano, finendola con la retorica delle risorse umane, che poi è indifferente a tutti gli strumenti concreti che le risorse umane davvero le aiutano aiutano a crescere e a lavorare bene. Del resto, era questo l'asse, il punto di partenza del Patto del 1993, 1993, ricordato dal presidente Romano Prodi, che poneva gli investimenti in formazione, ricerca ed innovazione a base di un confronto fra le parti sociali, non a somma zero, ma a somma positiva per il lavoro, le imprese e l'Italia. Mi pare che il DPEF abbia finalmente preso consapevolezza di questa verità e quindi spero che sia il preludio di una legge finanziaria che sappia mettere a disposizione le risorse politiche e culturali per approfondire, arricchire e dare senso alle stesse politiche di concertazione sociale. Il basso livello di sapere si supera innalzando i livelli di istruzione generale del Paese e premiando il merito e i talenti. Le due cose si possono fare insieme. È possibile una politica più inclusiva e di qualità. La scuola e l'università dell'autonomia hanno l'obiettivo fondamentale di costruire ed innalzare i livelli di istruzione e di sapere di massa e nello stesso tempo di valorizzare e premiare i talenti. Per farlo c'è bisogno di investire e di investire bene. La valutazione deve essere il naturale completamento dell'autonomia. Il Governo potrebbe, già dalla prossima finanziaria, raccogliendo le indicazioni che derivano economico-finanziaria in tema di università e ricerca darci un obiettivo preciso: portare gradualmente gli investimenti a livello dei Paesi europei più avanzati nella formazione superiore e nell'università e nel contempo aumentare la quota di risorse da assegnare tramite valutazione fino ad arrivare al 30 per cento del trasferimento. Perseguire gli obiettivi di Lisbona cambiando nel contempo la composizione interna della spesa ed aumentando gradualmente la quota dei trasferimenti tramite valutazione. Ci vorrà tempo, ma per arrivarci

i dati della ridotta mobilità sociale, secondo i quali l'istruzione, il fattore più potente di mobilità sociale oltre che di umano arricchimento, è così dispari. Il 71 per cento dei figli dei laureati ottiene iltitolo di studio liceale,

tanto che siamo autorizzati ad affermare che si pone una nuova questione meridionale, vale a dire una sorta di collasso dei tassi di rendimento e delle capacità di apprendimento dei giovani in consistenti aree del Sud. di programmazione economico-finanziaria siano di una particolare intensità riformatrice; esse vanno analizzate, interiorizzate e capite per il loro effetto sistemico. Molto è quello che il Governo ha fatto in questo anno e mezzo: l'obbligo, il potenziamento dei tecnici professionali, la maturità economico-finanziaria propone non è più la manutenzione, non è più la cosiddetta logica del cacciavite, non è più il molto e non è più la logica incrementale rispetto al già fatto, ma è l'altro,

cui offrire supporti, un diverso sistema contrattuale, l'incentivazione ed un altro modo di costruire i salari degli insegnanti. Quindi, ad un sistema scolastico rigido, economico-finanziaria fa un'altra offerta politica, cioè quella dell'autonomia, della responsabilità dei territori (che già fanno tanto), di un nuovo sistema di valutazione, dell'assunzione del ruolo del Titolo V della Costituzione italiana riformata, insieme ad una programmazione di lungo periodo di tutto quello che sta cambiando nella natalità, nei bambini immigrati e nell'età della gente che utilizzerà il sistema scolastico. Voglio, dunque, sottolineare

è chiaro: per ottenere l'obiettivo del pareggio, non è possibile accrescere la pressione fiscale perché si contraddirebbe l'obiettivo di rilancio della crescita e dello sviluppo; non è possibile ridurre la spesa in conto capitale perché si contraddirebbe l'obiettivo di rilancio e di sviluppo; non è possibile agire sulla spesa per interessi perché quest'ultima è determinata dal livello del debito e dai tassi di interesse fissati dal mercato.

anzi, ha aggiunto che, con i conti del DPEF, per ottenere quel risultato di pareggio di bilancio entro il 2011, senza alzare la pressione fiscale contributiva, senza ridurre la spesa in conto capitale, è necessario che la spesa corrente in rapporto al PIL si riduca da qui al 2011 di tre punti percentuali 2011 di tre punti percentuali di PIL. Noi crediamo che la proposta del Governo debba essere accolta e che sarebbe una novità importante se finalmente il Parlamento opportunamente aggiungesse al limite di saldo un limite di spesa pubblica corrente primaria, cioè al netto degli interessi. Crediamo che sia necessario disegnare un percorso che conduca a quell'obiettivo - il pareggio di bilancio - senza aumento della pressione fiscale e senza riduzione della spesa per investimenti che quindi sia necessario fissare nella risoluzione del DPEF un percorso che porti a quell'obiettivo. Con il presidente Dini, presenteremo un emendamento alla risoluzione di maggioranza, che, accogliendo la proposta del Governo, fissi il percorso per raggiungere quell'obiettivo.

ma crediamo che sia necessario uscire da questa discussione, in primo luogo, con l'innovazione fondamentale del limite alla spesa pubblica corrente primaria e, in secondo luogo, con un percorso che sia coerente con quanto il Governo ci ha chiesto per raggiungere il pareggio di bilancio, cioè una riduzione consistente da qui al 2011 della spesa corrente primaria. Pensiamo che questo potrebbe migliorare molto la qualità dell'aggiustamento di finanza pubblica che siamo chiamati a condurre. Pensiamo che questa sia la strada che può davvero aiutare il rilancio della crescita e dello sviluppo nel nostro Paese. Spero che il Governo voglia anzitutto tener fede a ciò che esso stesso ha chiesto al Parlamento, cioè l'inserimento del vincolo di spesa primaria corrente, e spero che il relatore voglia considerare con attenzione l'emendamento che ci apprestiamo a presentare.

nell'esprimere un giudizio di carattere generale e sostanzialmente positivo rispetto all'impianto del DPEF e un apprezzamento per la relazione svolta all'inizio dei nostri lavori dal senatore Ripamonti,

sociale, necessarie a portare il nostro Paese al livello dei Paesi più avanzati dell'Unione Europea. Si sottolinea, inoltre, come nel nostro Paese si registri un tasso di povertà sopra la media europea: persone non autosufficienti spesso a carico esclusivo delle famiglie, situazione abitativa critica e, soprattutto (un dato assolutamente sconcertante,

l'emergenza sociale non ha subito un'inversione di tendenza. È invece aumentato il numero delle persone che stanno vicine alla soglia di povertà ed è aumentato l'indebitamento delle famiglie,

continua ad essere uno dei più bassi in Europa e l'area della precarietà del lavoro e del sottosalario è aumentata,

Tale situazione non è certo imputabile alla politica di questo Governo, perché è frutto di scelte politiche che da oltre 15 anni hanno individuato nella sola questione del costo del lavoro, della precarietà e della flessibilità l'unico fattore sul quale intervenire,

e questo ha creato molte aspettative nei nostri elettori. Tali aspettative erano e restano ancora molto alte,

comunque dato un po' di respiro e sollievo, quanto meno alle pensioni più basse. L'accordo sulla revisione dello scalone, ha certo migliorato

rapporti di lavoro flessibili, che non significa precari, rispondano alle esigenze di flessibilità dell'impresa. Ci troviamo invece in una situazione per cui tutta la partita relativa alla precarietà ad oggi non è stata affrontata.

dopo l'ultima crisi di Governo - del superamento della cosiddetta legge n. 30 e quindi della messa in moto di un meccanismo che gradualmente porti al superamento della precarietà e limiti quella che oggi viene chiamata flessibilità vera,

se vogliamo recuperare il consenso dei nostri elettori, che ha avuto la caduta vertiginosa che ha avuto e che può ulteriormente aumentare e trasformarsi in

dall'affermazione del principio che il lavoro flessibile, proprio perché è lavoro precario, proprio perché pone il lavoratore in una condizione

modo, se vogliamo ridurre la piaga della precarietà del lavoro a *part time* bisogna far rientrare all'interno dei contratti la possibilità di accedere al *part time* secondo le causali e la limitazione del tempo di reiterazione.

per il superamento della precarietà all' interno della pubblica amministrazione, perché se non comincia lo Stato a dare l'esempio, diventa assolutamente difficile che l'esempio venga seguito dai datori di lavoro, che tendenzialmente non ne hanno mai abbastanza.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori. Il ministro dell'economia Padoa-Schioppa, in occasione di un' audizione in Commissione bicamerale per le questioni regionali, ha presentato alcuni numeri molto importanti circa la quota della spesa pubblica complessiva di competenza di Regioni ed enti locali. Voglio qui ricordare Regioni ed Enti locali gestiscono il 30 per cento della spesa corrente complessiva dello Stato. E questo naturalmente lo si deve ai numerosi servizi di loro stretta competenza che sono stati incrementati sia dalle cosiddette leggi Bassanini della fine degli anni '90 che dal nuovo Titolo V della Costituzione: Regioni ed enti locali sono, inoltre, titolari di ben il 60 per cento del complesso delle spese in conto capitale dello Stato. Quindi vuol dire che il 60 per cento degli investimenti complessivi della pubblica amministrazione passano attraverso il sistema delle Regioni e degli enti locali. Credo, quindi, sia molto importante, come la stessa Commissione bilancio del Senato ha riconosciuto, discutere ed affrontare preliminarmente alla legge finanziaria il tema del rapporto tra i i vari comparti di spesa, soprattutto distinguendo tra il livello centrale e quello locale e regionale. È stato anche approvato un documento che io credo importante, che andrebbe attuato, sulle nuove norme di formazione del bilancio, che prevede una preliminare discussione e, se possibile, elaborazione di un vero e proprio Patto almeno triennale di stabilità, rispetto al quale poi le leggi finanziarie annuali stabiliscono le varie quantità. Non può, quindi, sfuggire né al Governo né a noi parlamentari il fatto che il 5 luglio, quindi qualche settimana fa, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con un documento del proprio Comitato direttivo, abbia abbandonato di fatto tutti i tavoli di negoziazione, di discussione con il Governo, denunciando una situazione di totale insoddisfazione su tre punti fondamentali: l'uso dell'avanzo d'amministrazione da parte dei Comuni - nel decreto legge n. 81 c'è una soluzione molto parziale del problema il tema del Patto di stabilità che non consente di attuare gli investimenti programmati ed il tema dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale, il quale nonostante sia stato affrontato dal Governo con una proposta di legge in corso di esame, non vede però la soddisfazione dell'ANCI nel merito del testo presentato. Credo che questo sia un fatto istituzionale. Il Governo se ne deve fare carico e deve assolutamente creare le condizioni per ripristinare una normale e corretta dialettica istituzionale perché non c'è dubbio che i Comuni italiani sono parte integrante appunto della Repubblica, dello Stato. Da loro dipende grande parte della spesa pubblica ed è necessario coinvolgerli nella decisione circa le grandi scelte che attengono la spesa. economico-finanziaria, l'ANCI solleva un paio di questioni che sono molto rilevanti e che in parte accennavo or ora. Quella più rilevante è, secondo me, la questione relativa al Patto di stabilità. Non c'è dubbio: chi come me siede su questi banchi del Senato, nel corso degli ultimi cinque anni quando eravamo all'opposizione, ha fatto battaglie contro una certa interpretazione di Patto di stabilità, intesa in termini esclusivi di tetti di spesa. Si è passati ai saldi ma tutto questo non consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che sono risorse proprie dei Comuni, né consente tanto meno gli investimenti programmatici. È una cosa cui occorre porre rimedio. Infine, accennavo prima al tema dell'articolo 119 sul federalismo fiscale per il quale sarebbe necessario tener conto che la Costituzione prevede il finanziamento delle funzioni amministrative, laddove esse sono allocate. Questo è un principio fondamentale, che può aiutare anche a superare un conflitto in atto tra Comuni e Regioni su questo punto che, se se non trova soluzione, può dare solo luogo a fatti negativi. Invito, quindi, il Governo a tener conto di questi temi e il Parlamento, nel momento in cui approverà la risoluzione di approvazione del DPEF, a farsene carico, in modo tale che con la finanziaria del 2008 si ponga rimedio ad una situazione di conflitto istituzionale che non può assolutamente essere lasciata senza soluzione.

vorrei spendere qualche considerazione, anche un po' più politica, un po' più forse sopra le righe, rispetto a questo documento. Molti hanno sottolineato negli interventi che mi hanno preceduto alcuni aspetti un po' rinunciatari di questa manovra. Se noi paragoniamo questo documento a quello che è stato presentato lo scorso anno, notiamo un salto di qualità, perlomeno psicologico, verso il basso. Lo scorso anno avevamo una maggioranza un Esecutivo assolutamente arrembanti, che mettevano insieme un credo dirigista con l'adagio, che fu proprio di Bartali, che era tutto da rifare. Ma quell'impostazione si scontrò via via con un risultato già evidente in sede poi di manovra finanziaria successiva al DPEF, di errore, proprio di sbaglio interpretativo della realtà italiana e dell'eredità del Governo precedente e poi, più banalmente, di sbaglio clamoroso e con pochi precedenti sulle entrate. Oggi quella maggioranza è certamente più cauta,

dà l'idea di una maggiore prudenza ritrovata, di maggiore attenzione nel considerare le entrate, di una maggiore concretezza, purtuttavia si resta molto nel vago per ragioni che di qui a breve cercherò di rendere evidenti

tesoretto e alle spese, che si trovano al di fuori dei saldi di questa manovra. Sono spese che vengono elencate a parte perché non sono sorrette da norme di legge, ma sono spese

una serie di questioni per le quali il livello di esposizione è certo e a fronte delle quali parliamo di un diaframma da superare di circa 20 miliardi. Per non contare poi le ricadute ulteriori, il DPEF ce ne dà puntuale informazione, che riguardano l'aumento della spesa corrente per interessi, che viene prudenzialmente stimata, se non ricordo male, in 2,5 miliardi di euro in incremento (ma è appunto una stima ancora prudenziale). Tutto ciò dovrebbe trovare una risposta, che non è chiara nel DPEF, in una manovra che non dovrebbe comportare aumenti fiscali e dovrebbe portare a una riduzione di spese che non è ben chiara; è generalizzata: è un intento, un'aspirazione, ma non è ben chiaro dove andrebbe a cadere. perché tutto questo è politicamente debole e poco convincente? Per l'ottima ragione che un Governo che è nella condizione in cui si trova quello attualmente in carica ben difficilmente può procrastinare al 2011 qualsiasi cosa. Uno spostamento di obiettivi strategici a quella data per un Governo che secondo le persone più ottimiste è destinato ad essere in sella per i prossimi otto mesi è già di per se stesso un lancio della spugna.

sindacati, sono prive di qualsiasi fondamento, già smentite prima dell'approvazione del DPEF, se non mi sono ingannato venendo qui questa mattina leggendo sui muri della città, che l'accordo raggiunto dai sindacati, secondo autorevoli partiti non va bene e che la lotta continua. Evidentemente non credo che sia una lotta contro Alleanza Nazionale o Forza Italia, immagino che sia la lotta di alcuni partiti in Parlamento contro il Governo in carica per cambiare quell'accordo

nel modo che possiamo già misurare dalle prime reazioni che ci sono state, si accanisce non soltanto l'opposizione, non soltanto buona parte delle parti sociali, ma anche alcuni partiti, addirittura della maggioranza, che ne smentiscono parti rilevanti, in particolare quelle che riguardano in particolare quelle che riguardano l'accordo sulle pensioni. Insomma, autorevolissimi commentatori, all'unanimità, ciascuno per il suo verso, ciascuno dalla sua angolazione, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, l'Unione Europea convergono nel Europea convergono nel reperire le contraddizioni e le debolezze che in pochi minuti sto cercando di evocare all'attenzione dell'Aula. Il problema è quindi non di natura programmatica, ma di natura squisitamente politica. In qualche misura quello che è successo ieri in quest'Aula ne è la cartina di tornasole: la maggioranza ieri aveva i numeri, la tranquillità, la serenità - credo - per poter vincere tutte le votazioni senza alcun problema, soltanto che a questa maggioranza manca un elemento fondamentale, e cioè che quando dai banchi del Governo arriva la parola magica («Qual è il parere del Governo?», «Il parere del Governo è favorevole»), non scatta l'automatismo che, se il parere è favorevole, c'è una maggioranza che lo vota. Ora, questo elemento nel precedente DPEF era nascosto. Devo dire che il precedente DPEF, pur sbagliando completamente alcune previsioni in maniera grossolana, sembrava far trasparire la convinzione che questa maggioranza ritenesse le differenze al proprio interno non voglio dire una ricchezza, ma comunque un difetto, un *handicap* occultabile. Questo DPEF parla con chiarezza, invece, di come queste divisioni rendano sostanzialmente difficile, se non nullo, un ruolo di questo esecutivo ai fini di favorire la crescita del Paese in una congiuntura in cui alcune cose importanti potrebbero essere fatte facendo interventi strutturali sulla riduzione della spesa e cercando di cominciare a ragionare sulla riduzione della pressione fiscale e non si possono fare, per ragioni che - ripeto - sono tutte politiche, tutte interne alle contraddizioni di questa maggioranza. Va da sé qualora l'accordo sulle pensioni trovasse soprattutto in quest'Aula, che è quella dove è un po' più facile che accadano delle cose, elementi correttivi, tutto questo racconto finirebbe col ricadere su se stesso, nel senso che alla fine di questa discussione noi potremmo scoprire di avere approvato un DPEF sbagliato esattamente come era sbagliato quello dello scorso anno sulla previsione delle entrate, in questo caso sbagliato perché sconta un'idea che non è socialmente sostenibile per questa maggioranza, cioè quella di riformare le pensioni così come è le cose

ha raggiunto livelli che sono sconosciuti; bisogna risalire ai tempi in cui in questo Paese si votava per censo per trovare Governi più isolati e più distaccati dalla realtà sociale del Paese.

che è fondamentale: senza coesione sociale è impossibile perseguire qualsiasi tipo di obiettivo, non si può perseguire la competitività, non si può perseguire il contenimento della spesa, non si possono perseguire le politiche di risanamento. Anche su questo punto, credo che il passo che è stato fatto, buttando tra le gambe degli italiani alla vigilia dell'estate un accordo sulle pensioni che mette in difficoltà le stesse parti sociali che lo hanno firmato, chiunque ha visto (io non l'avevo visto, ma me lo hanno registrato e me lo hanno fatto vedere) quello che è successo davanti ai cancelli delle fabbriche, riportato dalle immagini televisive, dove solamente un sindacalista diceva che era a favore dell'accordo e tutti quelli che uscivano da Mirafiori si dichiaravano contrari (tutti, non i più politicizzati o i più scalmanati) ci dà la dimensione di come si stia, anche da questo punto di vista, perdendo la premessa necessaria a fare un Documento di programmazione economico-finanziaria condiviso e di effettivo rilancio. Quindi - e concludo davvero da questo punto di vista, al di là dei numeri sui quali qualcosa abbiamo detto in questi dieci minuti e molto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, al di là degli interrogativi che restano aperti sulle sulle coperture di spesa e sulle effettive capacità di questo esecutivo di comprimere la spesa pubblica, al di là delle importanti riflessioni sul debito che sono state poste al centro dell'attenzione di questo dibattito, il punto è squisitamente politico. Un Governo che nella percezione della sua stessa maggioranza, degli italiani, del suo elettorato oltre che della opposizione, che vive in questa aspirazione in qualsiasi democrazia parlamentare, ha i mesi contati, evidentemente ha qualche difficoltà ad intrattenere quest'Aula ed il Paese sulle politiche di rilancio complessivo dell'Italia e sulla capacità della nostra nazione di recuperare competitività sui mercati internazionali. È un fardello che diventa pesante perché ovviamente non è di questo che avrebbe bisogno il Paese in queste ore. il Documento di programmazione economico-finanziaria analizza la situazione economica del Paese mettendo in evidenza il fatto che l'Italia, anche grazie alla rigorosa manovra finanziaria dello scorso anno, sia uscita da una situazione di stagnazione economica e si sia avviata efficacemente sulla strada del risanamento dei conti pubblici.

È apprezzabile quanto è stato fatto nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, ma occorre ancora fare molto su questo terreno, anche per rimodulare e riequilibrare la pressione fiscale, ad esempio attraverso la tassazione delle rendite finanziarie o delle cosiddette pensioni d'oro. Il risanamento dei conti, dunque, non è stato accompagnato finora da un reale miglioramento delle condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini di questo Paese. Nello stesso DPEF si afferma che per far sì che il miglioramento della situazione economica italiana si traduca in un fenomeno strutturale consolidato è necessario che vengano avviate politiche che siano eque sotto il profilo sociale e sostenibili sul piano ambientale. allora dare seguito e concretizzare in precise scelte nella prossima manovra finanziaria quanto si afferma nel DPEF, ad esempio a proposito di piena e buona occupazione, attraverso decise azioni contro le forme precarie e precarizzanti del lavoro e della vita stessa; quando si parla di politiche per l'inclusione sociale e per la lotta alla povertà; quando si dice di voler investire nella ricerca e nell'innovazione e di voler rilanciare la scuola pubblica e l'università; quando si parla di politiche per il Mezzogiorno, stabilendo obiettivi misurabili e verificabili per i servizi essenziali, per il benessere e le prospettive delle comunità locali, ancora particolarmente inadeguati; quando si sottolinea l'impegno per una seria politica ambientale, a partire dal rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Relativamente a infrastrutture, mobilità e reti di telecomunicazioni, temi che l'8a Commissione ha analizzato puntualmente ed approfonditamente, è condivisibile quanto contenuto nel capitolo sulla mobilità in cui si ribadisce che l'obiettivo è quello di realizzare un sistema di trasporti sicuro, efficace e sostenibile; che è necessario stabilire principi guida per il soddisfacimento dell'interesse collettivo all'interno del Piano generale della mobilità, in cui si individuano azioni per il potenziamento di un modello di mobilità sostenibile, puntando sulla razionalizzazione della mobilità urbana, sul trasporto ferroviario, sulle vie del mare, sulla portualità, sulla logistica. Analogamente sono condivisibili, per quanto riguarda le reti di telecomunicazioni, le intenzioni di superare il *digital* *divide* soprattutto nelle aree marginali del Paese, migliorando il livello di penetrazione in termini di accesso alla banda larga e mettendo in atto azioni che assicurino l'universalità dell'accesso a Internet*,* incentivando anche le nuove tecnologie *wireless*. È importante che il Documento abbia ribadito la volontà di valorizzare l'infrastruttura fisica e tecnologica di 1.400 uffici postali, che potranno garantire anche nelle aree interne un'offerta di servizi pubblici tecnologicamente avanzati. In riferimento all'edilizia abitativa, è importante che il tema torni ad essere presente nell'agenda politica del Governo, definendo un programma nazionale sulle politiche abitative per incrementare il numero di alloggi a canone agevolato, di alloggi di proprietà per particolari categorie sociali, di alloggi di edilizia pubblica. Vorrei segnalare, però, l'incongruenza, già evidenziata in Commissione, tra le linee politiche relative alla mobilità e l'elenco delle opere infrastrutturali prioritarie dell'allegato infrastrutture. Riteniamo, infatti, che il Piano delle infrastrutture dovrebbe essere subordinato, consequenziale, al Piano della mobilità. Nel DPEF si ribadisce che le priorità infrastrutturali devono essere informate al soddisfacimento dell'interesse collettivo e inoltre che la valutazione per le scelte degli interventi prioritari deve basarsi sulla rigorosa applicazione dell'analisi costi-benefìci, coerentemente con le procedure di valutazione richieste dalla Comunità Europea. Nella prima parte dell'Allegato infrastrutture si sottolinea che l'individuazione delle priorità infrastrutturali dovrà essere coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, nel rispetto del Protocollo di Kyoto, della direttiva europea sulla qualità dell'aria e di quelle sui tetti nazionali delle emissioni inquinanti. La selezione strategica degli interventi dovrà poter incidere positivamente sul contrasto dei cambiamenti climatici che in Italia vede il comparto dei trasporti pesare per oltre un quarto del totale delle emissioni di gas serra. quindi lo stesso Allegato infrastrutture che segnala la necessità di un'ulteriore indicazione di priorità per le opere infrastrutturali contenute nel Documento, in coerenza con i principi di sostenibilità, riequilibrio modale, coesione sociale e tenendo conto delle risorse pubbliche e private effettivamente disponibili. Che coerenza c'è, però, se la maggior parte degli investimenti, cioè il 54 per cento, è per le strade e solo il 38 per cento Evidentemente, c'è bisogno di infrastrutture che assicurino il diritto ad una mobilità di qualità per tutti i cittadini ed anche per quelli delle aree interne, in particolare del Mezzogiorno e delle isole, cioè della Sicilia e della Sardegna. Proprio per questo bisogna operare delle scelte. Ci sono opere che forse non sono grandi per il giro d'affari, ma possono contribuire a migliorare realmente la qualità della vita delle persone: la messa in sicurezza delle strade, l'efficienza, la puntualità e la pulizia dei trasporti pubblici, città meno congestionate e meno inquinate sono davvero grandi obiettivi da raggiungere. Per queste ragioni siamo per il superamento della legge obiettivo; lo abbiamo scritto nel parere ed è scritto anche nel programma dell'Unione, perché perché è necessario ripristinare la corretta programmazione delle opere, reintroducendo il ricorso alle procedure di impatto ambientale. È altresì necessario individuare percorsi condivisi, democratici, partecipati con le istituzioni locali e con i cittadini che hanno tutto il diritto di non subire passivamente

dedicherò questi minuti a sottolineare un punto particolare, cioè il contributo che, nella logica del DPEF, hanno i fattori produttivi ed in particolare il lavoro (altri colleghi hanno parlato degli altri aspetti), per dire che questo DPEF non solo è in continuità con quello scorso, ma ha già fatto un prezzo di strada e non è affatto un libro dei sogni come qualcuno vuol dire. Il lavoro ha contribuito al primo dei pilastri di cui si parla nel DPEF, cioè al risanamento, perché fino a poco tempo fa si rilevava una crescita delle retribuzioni molto contenuta e, quindi, un sacrificio in vista di un bene, cioè il risanamento, che serve anche ai giovani perché toglie il peso dalle spalle.

trovato attuazione perché - questo non è stato detto - non solo è cresciuta all'occupazione quasi dell'uno per cento, ma a differenza del passato è aumentata la produttività del lavoro e in generale del nostro sistema, certo non ancora ai livelli europei ma per la prima volta in modo significativo;

Questi primi risultati, quindi la ripresa della crescita, dell'occupazione, della produttività, non sono solo frutto di fortuna internazionale, ma anche di alcuni provvedimenti già attuati e di altri in cantiere. Il fatto che in questi mesi abbiamo attuato alcune indicazioni in tema di regolarizzazione del lavoro, di emersione del sommerso, di alleggerimento del costo del lavoro sono tutte piccole indicazioni che portano a questo risultato. In proposito, faccio notare che l'entrata a regime della riduzione di tre punti del costo del lavoro (ci stiamo

Come si ottiene questo? Si ottiene ponendo in essere gli altri provvedimenti che nel DPEF sono indicati, alcuni dei quali sono già stati oggetto dell'accordo, raggiunto con qualche fatica, ma significativo,

ad una situazione pregiudicata dal precedente Governo. Ma sullo scalone è importante che questo giusto ammorbidimento venga coperto come è previsto per iscritto, perché se non lo fosse allora sì che avremmo effetti negativi sulla spesa e quindi anche sulla crescita. Gli altri provvedimenti, però, non hanno solo valore distributivo: le pensioni basse lo hanno, ma provvedimenti come, appunto, la riduzione del costo del lavoro, gli stessi ammortizzatori sociali che sono stati concordati hanno un effetto di di spinta per una crescita che si basi anche sulla ristrutturazione, sulla mobilità dei fattori produttivi. Si tratta quindi di uno strumento di cui avevamo bisogno. Abbiamo indicato un punto importante: dare soldi alla produttività e alla riduzione dei costi eccessivi dello straordinario, il che vuol dire garantire più soldi in busta paga ai lavoratori e produrre stimoli per l'impresa, con un doppio effetto virtuoso. Questi sono i tasselli concreti che servono

di approvazione ed è oggetto di un accordo sociale che deve reggere e poi, guardando più lontano, ci sono provvedimenti di più ampio respiro. Cosa manca al nostro motore per il lavoro, per essere a pieni giri? Mobilizzare la forza lavoro femminile. Qui si parla di un piano di sviluppo del lavoro femminile. Nelle nostre Commissioni sono incardinati due-tre disegni di legge sulla conciliazione e questo è il futuro. Segnalo, per finire, che gli obiettivi posti alla fine della legislatura, cioè del periodo considerato dal DPEF, sono ambiziosi: una crescita dell'occupazione al 61,5 per cento (quindi, un tasso di occupazione ambizioso) e una crescita

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011 presentato dal Governo desta, a mio avviso, talune perplessità. Ciò che mi rende maggiormente perplesso è il dover constatare che le conclusioni emerse dal dibattito svoltosi sulla politica fiscale e finanziaria, hanno trovato poco riscontro nel testo del Documento in esame. Per settimane e settimane abbiamo esaminato e criticato la politica fiscale e finanziaria fin qui adottata. Il Governo ha accolto molte delle nostre istanze, promettendoci di tener conto delle nostre preoccupazioni e di provvedere - visto l'andamento positivo delle entrate fiscali al cambiamento delle regole finora troppo punitive, soprattutto nei confronti delle imprese, ma anche delle famiglie. Esaminando il DPEF non ho, tuttavia, trovato la tanto auspicata e netta inversione di rotta nella politica fiscale e finanziaria; non vi è neanche traccia della tanto promessa sostanziale riduzione della pressione fiscale. Con grande rammarico ho potuto, addirittura, constatare che per le imprese sono previsti ulteriori e nuovi ostacoli burocratici. Non è così che si aiuta una ripresa economica fortunatamente in atto anche in Italia. Agli oneri burocratici già esistenti e gravanti sulle imprese, non ne andrebbero aggiunti nuovi. Essi vanno ridotti soprattutto se si ha a cuore il destino delle piccole e medie imprese. Alla luce di queste riflessioni, mi vedo costretto ad essere critico anche nei confronti della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione. È giusto contrastare l'abuso dei contratti flessibili per dare ai giovani maggiori certezze, altrimenti questi ultimi non potranno mai diventare autonomi ed economicamente indipendenti dai genitori. È inutile meravigliarsi del tasso di natalità in crescente diminuzione, se non si provvede a favorire la famiglia garantendo ai giovani le necessarie condizioni. Al tempo stesso, occorre, tuttavia, riconoscere che l'economia ha bisogno di flessibilità e questi contratti rappresentano spesso l'unico strumento valido per garantire una regolare assunzione del personale e contrastare il lavoro sommerso. Mi permetto di fare un esempio: se un albergatore ha bisogno, in via straordinaria, di ulteriore personale e deve impegnare magari per una o due giornate un lavoratore, magari uno studente o una casalinga ben felici di guadagnare qualche centinaio di euro, oggi ricorre al contratto di lavoro a chiamata. L'unica alternativa alla forma contrattuale, una volta abolita, è il lavoro in nero e non penso che ciò sia la soluzione auspicata dal Governo. In tutta Europa i processi di liberalizzazione vengono accompagnati da una maggiore flessibilità del mercato del lavoro. In Italia, invece, si vuole proseguire il processo di liberalizzazione, togliendo la flessibilità del lavoro. Questa, a mio avviso, è una forte contraddizione. Ho apprezzato molto l'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi sul DPEF. Non voglio ripetere le sue puntuali e precise osservazioni, ma soltanto rimarcare che i conti pubblici vanno tenuti sottocchio. Anziché pensare a nuove entrate dobbiamo contenere la spesa pubblica. Le scelte in materia previdenziale devono garantire la stabilità dei conti anche nel lungo periodo. Si possono ridurre le spese, per esempio, nel settore della pubblica della pubblica amministrazione, si possono, inoltre, tagliare i costi della politica, sia a livello nazionale che locale. Dopo anni di stagnazione, il Paese può finalmente tornare a crescere. Questa è una fase delicata ed è nostro compito dare al mondo economico il necessario sostegno. Mi auguro, quindi, che il Governo colga questa occasione per dare uno slancio al Paese, riducendo la pressione fiscale, adottando una politica di liberalizzazioni accompagnata accompagnata da maggiore flessibilità del lavoro, mantenendo sempre come obiettivo il risanamento dei conti pubblici. La dichiarazione di oggi del vice ministro Visco, che promette una riduzione della pressione fiscale sia per le imprese che per le famiglie a partire dalla prossima legge finanziaria, mi rende fiducioso in tal senso. Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, l'obiettivo politico di fondo del programma elettorale dell'Unione, condiviso non sole dalle forze politiche ma sostenuto dall'elettorato, è che gli obiettivi di crescita e di risanamento finanziario devono essere socialmente equi ed ambientalmente sostenibili. Lavoro, diritti e crescita camminano insieme. L'obiettivo rinviava a quell'economia della riproduzione sociale i cui tratti sono stati delineati dalla contro-Conferenza di Nairobi, passando per Pechino e Huairou, dalle economiste femministe e dalle rappresentanti delle organizzazioni non governative di ogni parte del mondo, di ogni parte del mondo, che ancora stenta ad affermarsi nelle istituzione economiche mondiali. C'è un sapere, maturato nell'esperienza quotidiana delle donne e degli uomini. Il presupposto dello sviluppo, di ogni sviluppo o comunque lo si voglia aggettivare - ne ho sentiti tanti di aggettivi nel corso della seduta odierna- è lo sviluppo umano e le sue determinanti sono il reddito, l'istruzione e la salute, in particolare delle donne. Non si tratta di questioni specifiche o di aspetti settoriali, ma di elementi strutturali per un'economia che parli alla cittadinanza (pólis) e alla democrazia (demos) e non solo alle cittadelle finanziarie. Questo ha fatto la differenza nel programma dell'Unione e su questo cambio di passo dovremo misurarci con la finanziaria. La salute, in particolare, è un bene inalienabile per le donne e per gli uomini, fondamentale alle loro relazioni, ed è un investimento sul futuro del Paese. Non è un capitolo di spesa da contenere o da comprimere. Lo dichiara e lo riconosce l'OMS, a differenza della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, che però hanno preso il suo posto nel definire gli indici dello sviluppo e tuttavia, sulle indicazioni dell'OMS si è fondato il programma dell'Unione e su di esso occorre investire riconoscendo che mentre la spesa sanitaria, secondo i dati dell'OCSE, è ancora sotto la media dei Paesi europei, sia in termini di livello che di tassi di crescita, il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per tutti e per tutte e su tutto il territorio nazionale è insufficiente. Per questo la sfida decisiva resta l'obiettivo del programma dell'Unione: adeguare il Fondo sanitario nazionale per dare garanzia piena in tutto il Paese di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche nella previsione di un loro progressivo, necessario allargamento a partire dalle cure odontoiatriche. Nello stesso tempo, va portato a consapevolezza che precarietà - la precarietà del lavoro ma anche quella generalizzata delle condizioni di vita che ne deriva - e salute sono elementi tra loro in contraddizione e lo sono qui ed ora. Questa contraddizione irrisolta peserà non solo sulle nuove generazioni, ma sulla società che si sta costruendo. Si tratta allora di segnare con questo tratto l'azione di Governo nella prossima finanziaria

di lavoratori e lavoratrici poveri, collegata alla precarizzazione dei processi di lavoro e alla perdita reale di potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Bisogna affrontare qui e oggi, non per le future generazioni (lo dico a beneficio del senatore Del Pennino,

cento non può sostenere una spesa straordinaria di 600 euro e una spesa del genere è quasi all'ordine del giorno se non si interviene rifinanziando il fondo sanitarionazionale. Ci è stata consegnata una questione sociale sulla casa, con affitti che divorano salari e pensioni. Vi è poi una questione sociale in relazione all'insufficienza dei servizi di assistenza alle persone non autosufficienti, di servizi educativi per la prima infanzia, di servizi scolastici per tutte e per tutti. C'è un grande bacino di salute e benessere da guadagnare. Ce lo eravamo guadagnati negli anni passati e lo verifichiamo oggi grazie alla crescita dell'aspettativa di vita e anche grazie ad un servizio sanitario nazionale universalistico. È questo il terreno sul quale va tenuta ferma la barra del programma dell'Unione perché nei Paesi in cui ci si compra ognuno per sé i servizi i cui si ha bisogno non cresce il Paese, non c'è sviluppo, non c'è economia possibile.

aver deciso per l'anno prossimo di qualificare l'offerta e quindi di fare una politica di sviluppo finanziandola con un taglio lineare per 21 miliardi di euro, senza procedere pertanto ad una manovra aggiuntiva; nello

come si può avere fiducia in un Governo che si è dilungato ad affermare che avrebbe tagliato le tasse e che poi, soltanto qualche mese dopo avere riempito tutti i giornali, le trasmissioni televisive e le Aule parlamentari sostenendo che le tasse sarebbero calate, che la pressione fiscale sarebbe diminuita e che l'IRPEF avrebbe riguardato tutti quelli al di sopra o

di credere che possa dare lo sviluppo che il Paese si attende di poter ricevere con un'azione di Governo e con una programmazione che ha un'assoluta impossibilità

sostanzialmente verificato, cioè un inusitato aumento della pressione fiscale e contemporaneamente uno sviluppo che non coglie la contingenza internazionale, che in altro modo, invece, avrebbe potuto essere colta.

che stiamo discutendo è connotato da caratteri di particolare innovatività ed è in coerenza con la politica economica e finanziaria inaugurata con il DPEF di legislatura dello scorso anno. Le innovazioni discendono, a mio modo di vedere, dall'accelerazione su determinati obiettivi resa possibile dall'indubbio successo della manovra dello scorso anno, che - come è a noi tutti noto ha consentito di ottenere il necessario risanamento finanziario, andando oltre gli obiettivi programmatici fissati, in un quadro di crescita dell'economia e di primi interventi, pur se insufficienti, per conseguire più equità sociale. Il quadro delineato con il Documento programmatico di cui stiamo discutendo e i dati di finanza pubblica e di andamento dell'economia consentono di affermare che la prossima manovra si muoverà e potrà muoversi entro un perimetro segnato da alcuni punti certi. luogo, non è necessaria, come si è detto in quest'Aula e come ha riferito puntualmente il relatore, dopo tanti anni, una manovra correttiva, perché essa è stimata in circa 7,5 miliardi ed è già inglobata nei tendenziali, il che costituisce uno straordinario successo del Governo e della maggioranza, che possiamo a ragione rivendicare. In secondo luogo, la pressione fiscale non deve salire ulteriormente, anzi, come prevede il DPEF, possibilmente dovrà scendere. In terzo luogo, l'indicazione oltre i tendenziali delle previsioni tassonomiche contenute nel Documento, oltre a costituire un'indubbia operazione verità, che consente di disegnare l'orizzonte degli interventi obbligatori, necessari, opportuni o anche solo eventuali, costituisce il limite massimo della manovra, limite che auspico non venga raggiunto. Ciò in quanto - e vengo al quarto punto - le spese devono essere coperte con la riqualificazione e la riduzione di altre spese. È questa la sfida nuova che il Governo affida a sé stesso e al Parlamento, su cui si misurerà l'efficacia e la fattibilità della manovra. Il poco tempo a disposizione non mi consente ovviamente di entrare nel merito di questi e di altri punti. D'altronde, condivido appieno le indicazioni Mi limiterò soltanto a formulare due osservazioni, anche per confutare lo scetticismo da ultimo manifestato dal senatore Ferrara, la critica, l'unica teoricamente proponibile, circa il carattere asseritamente velleitario e irrealistico dell'impostazione sul punto del DPEF, ovvero che l'obiettivo di finanziare gli interventi ipotizzati (11, 13, 15 o 21 miliardi, si vedrà) solo agendo sulla leva della spesa, in particolare su quella primaria, non sarebbe conseguibile. Che l'obiettivo sia ambizioso è fuori discussione. Che la rigidità della spesa pubblica abbia nel passato consentito limitate operazioni è altrettanto noto. Rammento al riguardo l'insuccesso diffuso delle politiche dei tagli lineari o anche del meccanismo degli accantonamenti, previsto dal comma 507 dell'ultima finanziaria. Senonché, proprio l'insegnamento che ci proviene da tali inefficaci politiche può farci individuare la via da seguire, che il Governo, con la riclassificazione del bilancio e la *spending review* ha già imboccato, cioè quella di incidere in profondità sulle cause generatrici della spesa, quindi sulla legislazione vigente, e sulla qualità della stessa, nel senso di abbandonare programmi e obiettivi non più prioritari per privilegiarne altri. Numerosi possono essere gli esempi: in primo luogo, la tanto dibattuta questione dei costi della politica, quale fonte di finanziamento di altre spese.

la pressione fiscale, ma per raggiungere obiettivi di equità e di crescita. Infine, il Patto di stabilità interno

Comunico agli onorevoli colleghi, come già anticipato per le vie brevi ai Gruppi, che, al fine di rispettare i tempi previsti dal calendario, la seduta antimeridiana di domani è anticipata alle ore 9.

attiene perfettamente al caso in questione e che recita così: «Il lupo dalla mala coscienza come opera pensa». Immagino che il senatore D'Onofrio abbia rivolto quelle espressioni all'Aula, sollecitando applausi a scena aperta - mi si dice - per questa

possono in qualche modo avere irrobustito, non dico certo un partito democratico come l'UDC, ma la sua sfera di consenso personale. Questa prassi non ci appartiene e mi fa molto sorridere quando il senatore D'Onofrio fa riferimento alle sue battaglie per la Sicilia, per il Mezzogiorno, che non le ha mai ridotte a vili mercanteggiamenti. È noto che neanche il Movimento per l'Autonomia agisce per vili mercanteggiamenti, ma ha nella sua ragione costitutiva l'impegno per la sua terra. In questa volgare illazione del presidente D'Onofrio vi è poi un'offesa gravissima al Capo del Governo: del Governo: immaginare che un uomo certamente criticabile per la sua azione di Governo, ma moralmente irreprensibile come il Presidente Prodi possa aver in qualche modo contrattato l'assenza di un parlamentare dall'Aula in cambio di un finanziamento,

debba approfittare dell'autorevolezza della funzione di Capogruppo parlamentare perché, in condizioni di vantaggio come quelle di questa mattina, si possono arrecare danno e dispregio non soltanto al parlamentare (in questo caso si tratta del sottoscritto, oggetto di questa volgare illazione), ma anche all'istituzione, perché all'istituzione, perché immaginare questo tipo di scambio volgare è davvero un atto di offesa al Parlamento e alla sua attività. Per quanto mi riguarda, la mia assenza dall'Aula, che ho ampiamente motivato alla stampa ed alla stampa ed anche al mio Gruppo, era legata alla concomitanza già preannunciata di impegni politici molto rilevanti che non mi hanno consentito di essere presente in una serie di votazioni per le quali non ero in alcun modo decisivo, perché, da quanto risulta dai risultati ufficiali ufficiali delle votazioni elettroniche, non vi è stata mai, in alcuna occasione, la possibilità per l'opposizione di mettere in minoranza la maggioranza, visto che lo scarto minimo è stato di circa sei voti. Si tratta, quindi, davvero di una grave ed ingiustificata offesa.